Signori senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero di vicinanza e cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici della senatrice Carla Nespolo, scomparsa domenica scorsa dopo una lunga malattia. Donna di vivace intelligenza e forti principi morali, Carla Nespolo è stata tra le principali protagoniste di tante battaglie sociali, culturali e legislative della nostra storia. Nata negli anni più bui e drammatici del secondo conflitto mondiale, in un'Italia divisa dall'odio e dalla violenza fratricida, Carla Nespolo non aveva fatto la resistenza ma ne aveva ereditato lo spirito, insieme a un amore incondizionato per quegli ideali di libertà e di democrazia che sono il cuore della nostra Costituzione. Su quegli ideali ha costruito la sua vita e la sua opera prima come insegnante e poi come donna di valore al servizio dei cittadini e delle istituzioni. Un percorso iniziato giovanissima come consigliere provinciale ad Alessandria a soli ventisette anni e culminato con la sua elezione prima alla Camera dei deputati e poi al Senato della Repubblica. Nel corso dei suoi quattro mandati parlamentari Carla Nespolo è stata firmataria e relatrice di importanti disegni di legge in materia di lavoro, istruzione, diritti delle donne, tutela dell'ambiente e dei territori; un impegno politico vissuto sempre con passione, coerenza, instancabile fedeltà ai suoi ideali, intelligenza e non comune apertura al dialogo e al confronto democratico, quella stessa passione che ha contraddistinto la sua azione all'interno dell'Associazione nazionale partigiani italiani di cui è stata prima presidente donna. Sempre presente a ogni manifestazione ed ad ogni anniversario, fino a quando la malattia glielo ha concesso, non ha mai smesso di difendere, raccontare e tramandare, soprattutto alle più giovani generazioni, l'eredità storica e culturale della Resistenza. Con Carla Nespolo ci lascia una donna straordinaria, l'esempio di uno spirito combattivo e determinato a dimostrare sempre il valore inestimabile di un Paese veramente libero da soprusi, prevaricazioni e violenze. In ricordo della senatrice Carla Nespolo invito pertanto l'Aula ad osservare un minuto di silenzio.

Signor Presidente, deputata dal 1976 al 1983 e senatrice dal 1983 al 1992, Carla Nespolo è stata presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia negli ultimi tre anni, la prima presidente donna, la prima non partigiana. Come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con Carla Nespolo perdiamo un'appassionata testimone ed una fervida sostenitrice dei valori della Costituzione. Da insegnante iniziò la sua opera di contrasto educativo e culturale a ogni forma di violenza e razzismo, proseguita poi nell'impegno parlamentare e quindi nella guida dell'ANPI. Per ragioni anagrafiche Carla Nespolo non aveva combattuto la Resistenza, ma era senza dubbio partigiana nelle idee e negli ideali, una profonda conoscitrice della storia e del suo valore. Anche questa sua passione spiega l'intransigente contrasto alla xenofobia. In un'intervista a Repubblica del 21 febbraio del 2018 aveva dichiarato: «Una cosa deve essere chiara: il fascismo trova il suo *humus* culturale nel razzismo. Le due cose vanno combattute insieme: dire ai poveri che i loro nemici sono i più poveri è la cosa più antidemocratica e ingiusta che si possa fare». C'è chi potrebbe chiedersi cosa serva oggi, a distanza di settantacinque anni dalla Liberazione, un'associazione di partigiani come quella presieduta da Carla Nespolo fino alla morte. Oltre che a combattere la malerba del fascismo, è Carla Nespolo stessa che ci dà il senso ed il valore di questa presenza ancora oggi. Durante i terribili venti mesi di guerra, i partigiani hanno sperimentato la forza dell'unità e sono riusciti a stare insieme, pur venendo da mondi diversi. Serve questo per rendere un Paese libero e democratico. Mantenere viva la memoria di quell'impegno e di quel sacrificio che sta alle fondamenta stesse della nascita della nostra Repubblica e della scrittura della nostra Costituzione è un dovere civico e politico importante. Carla Nespolo per prima lo ha fatto senza avere direttamente vissuto l'impegno nella Resistenza. Oggi il testimone della memoria e della lotta ad ogni fascismo deve passare a qualcuno di più giovane, che si farà nuovo testimone per tutti. nazionale partigiani d'Italia e dei suoi valori di democrazia non un reliquiario da onorare, ma un'esperienza a servizio di tutti per continuare a costruire il futuro. Ciao Carla. Ciao comandante. Bella, ciao.

Signor Presidente, ringrazio per l'occasione che viene offerta all'Assemblea per fare quella che io penso non possa che essere una doppia commemorazione. Da un lato, infatti, ricordiamo la figura di Carla Nespolo nella funzione che ha esercitato tanto più e soprattutto nella fase finale della sua esistenza, senza togliere nulla alla biografia importante che lei stessa, Presidente, ricordava e cioè quella di essere stata prima donna a capo di una grande organizzazione, anche molto complessa. In molti non conoscono infatti le dinamiche interne dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Prima donna a capo di un'organizzazione così importante e così complessa, ha svolto la sua funzione con grande determinazione, con caparbietà e anche con molta sensibilità, come quella che solo una donna può portare dentro un contesto di quel genere. Chi l'ha frequentata, chi ha avuto questo privilegio nei mesi più difficili della sua esistenza, prima che Carla si spegnesse, può raccontarci e ci ha raccontato di quanto fosse forte la sua determinazione nel portare avanti l'esercizio della sua funzione fino all'ultimo minuto disponibile e fino all'ultima risorsa fisica disponibile. Smuraglia, presidente emerito dell'Associazione, racconta di quando recentemente Carla lo chiamò nel cuore della notte perché assillata dal fatto che bisognasse ragionare e assumere una posizione su una vicenda politica. Carla Nespolo era questo e interpretava la sua funzione in questo senso, in un rapporto vivo con la società italiana e con il mondo dell'associazionismo, soprattutto non si è mai sottratta e non ha mai sottratto la sua associazione alle partite importanti della politica italiana, assumendo di volta in volta la posizione che lei riteneva fosse quella giusta, cioè quella di stare dalla parte della Costituzione e in difesa dei suoi valori. Carla Nespolo è stata tutto questo. in questi pochi minuti che ci vengono offerti c'è però un ulteriore significato di questa commemorazione che naturalmente vive in ragione del ricordo e della memoria di Carla Nespolo. L'occasione che noi dobbiamo darci e che soprattutto dobbiamo fornire al Paese in una discussione che va aumentata di scala, nel dibattito pubblico, deve ruotare attorno ad una domanda: cosa vuol dire essere antifascisti nell'Italia di oggi? Questo era un assillo di Carla Nespolo, così come lo è stato di tutti i presidenti dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia che l'hanno preceduta. due nemici che dobbiamo contrastare, al di là dell'appartenenza ai campi politici. Da un lato, una sorta di revisionismo strisciante, che esiste nel nostro Paese, più o meno esplicito, e che confonde in modo truffaldino la pietà che dobbiamo avere per i morti, tutti, e le vittime, tutte, con l'idea però che dobbiamo preservare e conservare, secondo la quale in ogni passaggio della storia c'è chi si siede dalla parte della ragione e chi invece decide deliberatamente di di stare da un'altra parte. Questo è un punto importante che va conservato e che deve far parte del patrimonio condiviso di un'intera comunità e di un intero Paese. C'è però un secondo nemico più subdolo, e su questo Carla ha combattuto ed ha esercitato la sua funzione in nome di questo contrasto. E cioè l'idea che non c'è soltanto una pagina della storia buia di questo Paese che richiama alla alla vicenda del fascismo, poiché il fascismo di ritorno non ha bisogno di divise per ripresentarsi nella storia, ma entra nelle pieghe della società in modo più insidioso e subdolo perché ha un volto diverso: quello del sopruso, della violenza, della negazione delle differenze, del razzismo, del contrasto al valore assoluto, che è quello della pace. Spesso dimentichiamo questa parola anche nelle nostre discussioni e quanto sia importante. Qui c'è la lezione di una figura importante come quella di Carla Nespolo, cioè l'idea che i valori della Resistenza e dell'antifascismo sono i valori delle nostre radici costituzionali e non sono relegabili semplicemente a una pagina di storia, ma devono vivere il rapporto con la società. In questo senso è molto importante la sottolineatura che ha fatto il collega che mi ha preceduto, perché è un passaggio inedito, ma fondamentale. Carla non era una partigiana in senso storico; non ha partecipato alla Resistenza, non fosse altro che per ragioni anagrafiche, ma la scelta dell'ANPI è caduta sulla sua figura anche in ragione del fatto che non fosse una partigiana in senso storico. Ma Carla partigiana lo era, perché sapeva da che parte stare; sapeva che doveva stare dalla parte della Costituzione e in questo senso penso debba essere ricordata, appunto, come una partigiana. Perché una persona che lavora e combatte nel segno della libertà muore anche per la libertà come ogni partigiano. Grazie, Carla, per quello che hai fatto. Ci mancherai.

Signor Presidente, Antonio Gramsci ha scritto: «Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani». Carla Nespolo non ha fatto la Resistenza, ma ha vissuto intensamente e politicamente; ha dimostrato cosa significa essere partigiani per le libertà, per la Costituzione. Per questo è diventata presidente dell'ANPI; prima donna, primo presidente che non ha fatto la Resistenza. Il nostro ricordo è per la sua intensa e autentica passione civile.

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, «combattente» è l'aggettivo più ricorrente nel ricordare Carla Nespolo in questi giorni. Voglio anch'io adoperarlo per la cifra della sua vita e del suo impegno politico, istituzionale e civico. Carla Nespolo se n'è andata a settantasette anni, dopo una lunga attività politica, svolta dentro e fuori le istituzioni, spesa ininterrottamente per rendere più robusta la coscienza democratica, più salde le istituzioni, più forte l'impegno nel miglioramento della società nazionale, che, per lei e la sua parte politica, significava diritti dei lavoratori, giustizia sociale, lotta contro ogni forma di discriminazione, economica e di genere. Parlamentare del Partito Comunista Italiano e del PDS, eletta in Piemonte, declinò il suo lavoro alla Camera, prima, e al Senato, poi, occupandosi di riforma della scuola secondaria, di emittenza radiotelevisiva, di ambiente e dei problemi di emancipazione delle donne. Combattente, dunque; prima donna - è stato detto - eletta presidente dell'ANPI e prima presidente a non aver partecipato direttamente, per motivi anagrafici, alla Resistenza. Ma proprio per questo importante la sua esperienza e il lavoro che ha fatto come ponte, come generazione ponte tra un prima e un dopo. elementi che hanno connotato il suo impegno nell'ANPI. Penso all'allestimento del Memoriale della Resistenza, un giacimento di memoria collettiva; ma penso soprattutto a come ha inteso essere dirigente dell'ANPI. Luciana Castellina l'ha definita: «Una grande partigiana dell'epoca presente», una combattente che ha interpretato il suo ruolo come impegno a schierarsi da una parte e che si è battuta molto per le celebrazioni del 25 aprile, fino alla fine. Voglio citare quanto disse a proposito della memoria: l'ANPI «serve per continuare una memoria che non è retorica, ma lotta per la costruzione di un Paese migliore». ricominciare dalla Costituzione vuol dire esattamente non ricominciare come prima. Già, perché il collegamento tra la lotta di liberazione e la Costituzione è stata la cifra del suo impegno politico e del messaggio che ha inteso sostenere, diramare e trasmettere alle generazioni di oggi e di domani. Combattente contro ogni forma di discriminazione e di razzismo, perché, come è stato detto e come lei ha affermato più volte, ha ritenuto e affermato con forza che il razzismo è alla base del del fascismo di ritorno. Combattente, non ha avuto paura e timore di schierarsi, anche con battaglie che potevano essere solitarie all'inizio, ma che, grazie al suo coraggio, non lo sono state; in prima fila per mobilitarsi contro i fatti di Macerata, per richiamare una responsabilità civica e una mobilitazione di popolo contro ogni tipo di paura e per difendere i valori della nostra Costituzione. Combattente per mettere fuori legge comunque ogni forma di ricostruzione dei partiti neofascisti e neonazisti. Combattente, però, anche per un altro aspetto, quanto mai attuale, che ha connotato quella generazione di ieri e di oggi che ha costruito la democrazia repubblicana nel nostro Paese. Combattente per l'unità, l'unità repubblicana. Non posso dimenticare, avendo partecipato con lei a una manifestazione istituzionale del 25 aprile, la sua irritazione per uno degli interventi che ebbero luogo quella mattina, di aperta polemica politica in un momento che doveva essere istituzionale - e non neutro - per questo motivo. Combattente per l'unità, perché l'antifascismo è la connotazione della nostra unità repubblicana. Combattente per le donne. La Resistenza non è stata solo maschile - lo ha detto più volte - e non è stata solo armata: le staffette, le gappiste sono state donne e sono state fondamentali e le donne hanno animato gli scioperi scioperi insurrezionali fatti in quel periodo. Intervenne nel 1985 sulla ratifica della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York, e denunciò il ritardo del nostro Paese. Disse che le leggi che hanno segnato la storia di milioni di donne nel nostro Paese hanno contemporaneamente segnato il cammino e lo sviluppo della democrazia italiana per tutti, uomini e donne. Signor Presidente, La Costituzione, la libertà, l'unità dell'Europa e l'apertura al mondo sono stati gli elementi costitutivi e ispiratori dell'impronta che Carla Nespolo ha voluto accentuare per l'Associazione che ha presieduto. Un esempio che ci spinge a lavorare per un Paese che trovi oggi la forza e l'unità per superare un difficile momento della sua storia. Cito ancora Carla: «La capacità di progettare un mondo migliore partendo da una storia tragica è una cosa che possiamo imparare dalla lotta partigiana».

che Carla ha svolto nei decenni, per amore del nostro Paese e delle generazioni di oggi e di domani. Ai suoi familiari, all'ANPI, ai suoi amici e alla città vanno il cordoglio e l'affetto del Gruppo PD del Senato. ha militato con quella che è stata la sua parte politica, oggi salutiamo una compagna coraggiosa, battagliera e coerente con i suoi ideali. Per chi ha condiviso allora con lei l'impegno istituzionale e che oggi rappresenta il Parlamento, salutiamo una testimonianza della politica vissuta come servizio e come impegno per il bene comune. Per i cittadini, tutti e soprattutto per quelli più giovani, salutiamo una patriota della Costituzione repubblicana, cifra identitaria che unisce e rappresenta un intero popolo.

Signor Presidente, unendomi, anche a nome del Gruppo Forza Italia, all'espressione di cordoglio per la scomparsa di Carla Nespolo, anch'io voglio ricordare l'impegno di questa donna nell'Italia repubblicana e del postguerra e il suo ruolo di presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia

ma per tutti coloro che si riconoscono nei valori della Resistenza, dalla quale sono nate la nostra Repubblica e la nostra Costituzione. Figlia di un partigiano delle Langhe e nipote del comandante Amino Pizzorno, com'è stato detto, Carla era una combattente e ha conosciuto tutte le atrocità del del ventennio fascista. È stata una combattente anche perché, fino all'ultimo dei suoi giorni, ha continuato a manifestare, anche da un letto d'ospedale, tutto il suo impegno a favore della libertà e della giustizia in difesa degli ultimi, quelli che lei considerava gli oppressi della nostra quotidianità, stando sempre al fianco di coloro che non rinunciano al sogno di un Paese più giusto, più solidale e più eguale. pedagogista, senatrice prima del Partito Comunista e poi del Partito Democratico della Sinistra, ma soprattutto una donna capace di rivendicare sempre e in ogni luogo qualunque battaglia che negli ultimi cinquant'anni sia servita a cambiare la cultura conservatrice di questo Paese. Non è un caso, dunque, che sia stata proprio lei la prima donna ad assumere il ruolo di presidente dell'ANPI, generando, peraltro, una grande attenzione da parte delle nuove generazioni per questa gloriosa associazione. Quando parliamo della Resistenza ai giovani - diceva Carla Nespolo - non dobbiamo farlo come se stessimo raccontando una stagione della nostalgia, ma parlando del loro futuro, perché questo è la Resistenza: il sacrificio di uomini e donne massacrati in nome dell'ideologia nazifascista, che ha reso possibile coltivare il seme prezioso della democrazia e che ha segnato uno spartiacque tra due idee del mondo, tra chi lotta per la libertà e chi per la sua negazione. La democrazia per tutti, anche per i vinti di allora, e per tutti la libertà e l'uguaglianza, senza discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche: questo era il sogno dei partigiani, che viveva e vive nella volontà di cambiare il mondo e che Carla Nespolo incarnava orgogliosamente. Essere antifascisti oggi - diceva significa essere contro il razzismo e contro chi approfitta anche della crisi sociale per far regredire politicamente, culturalmente e moralmente il nostro Paese; questi, troppo spesso fatti per perseguire facili ed effimeri consensi elettorali e che denotano una deriva valoriale rispetto alla quale lei, insieme all'ANPI, ha continuato a resistere come sentinella della nostra democrazia. In questo impegno una forza politica giovane come il MoVimento 5 Stelle si riconosce pienamente con i suoi militanti e i suoi rappresentanti in Parlamento, consapevole, soprattutto in una fase di così acuta difficoltà per i cittadini, che le istituzioni ereditate dalla Resistenza vanno difese ogni giorno nel Paese e in Parlamento, custodendo il loro corretto funzionamento e i delicati equilibri tra i poteri repubblicani. Tali equilibri proprio oggi, con il Paese appunto alle prese con un'emergenza economico-sociale senza precedenti e che ci chiama tutti a uno sforzo unitario per la ricostruzione pari a quello che i Costituenti seppero produrre negli anni drammatici del Dopoguerra, comportano un religioso rispetto dei ruoli, a cui il presidente della Repubblica Mattarella ci invita, affinché il Governo possa fare il suo lavoro e le Camere vigilare, legiferare e accompagnare questo sforzo lealmente, evitando che i loro più illustri rappresentanti si abbandonino a inopportune invasioni di campo. è la lealtà repubblicana cui noi, eredi e beneficiari dell'enorme e nobile lascito della Resistenza, siamo chiamati a praticare rigorosamente negli interessi di tutti i cittadini democratici di questo Paese, anche e soprattutto oggi, in nome di

voglio anch'io ricordare Carla Nespolo per tre brevi profili. In primo luogo, voglio ricordare la sua lunga attività politica, che è stata sempre saldamente radicata in profonde convinzioni morali, in ideali e in principi per cui si è battuta con una profonda, inscalfibile e rara coerenza. Voglio poi ricordare Carla Nespolo come donna, non solo impegnata in prima linea in tante battaglie per i diritti delle donne, ma anche perché la sua stessa vita è stata una testimonianza, direi un manifesto, contro tutti gli stereotipi di genere, tanto radicati - come sappiamo o non sappiamo - nel mondo politico, come dimostra anche, da ultimo, il suo essere stata la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente dell'ANPI. Vorrei infine ricordare e prendere a memoria come eredità spirituale di Carla Nespolo, per tutti noi, queste sue parole: «Il senso stesso del nostro impegno come ANPI, ma più in generale come democratici e antifascisti, è quello di combattere l'indifferenza».

quando scompare qualche senatore o qualche personaggio degno di essere particolarmente ricordato, come in questo caso Carla Nespoli, facciamo solo notare - e ci spiace che, anche in occasione del ricordo di una persona scomparsa, ci siano Gruppi politici che utilizzano questa occasione per attaccare strumentalmente partiti presenti o idee che sono rappresentate nel nostro Paese. Lo trovo davvero di uno squallore incredibile.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio ed è costituito da due parti: il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa. Il rendiconto è corredato dal rendiconto economico e da una relazione illustrativa, l'ecorendiconto dello Stato, che illustra le risultanze delle spese ambientali delle amministrazioni centrali dello Stato, ovvero delle spese aventi per finalità la protezione dell'ambiente e l'uso e la gestione delle risorse naturali. Venendo alle risultanze contabili, la gestione di competenza ha fatto conseguire, nel 2019, il miglioramento di tutti i saldi rispetto alle previsioni definitive, nonché rispetto ai risultati differenziali registrati nell'esercizio precedente.

In particolare, il saldo netto da finanziare, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, si attesta in campo positivo, di circa 2,3 miliardi di euro, ossia lo 0,1 per cento del PIL, con un miglioramento di quasi 22,3 miliardi di euro rispetto al saldo registrato nel 2018, che si era attestato a meno 20 miliardi. Il miglioramento del saldo è di circa 59,7 miliardi di euro, il 104 per cento, se confrontato con le previsioni definitive del 2019, che che indicavano ancora un valore negativo del saldo di meno 57,4 miliardi. Il risultato dà luogo a un accreditamento netto in controtendenza rispetto agli anni precedenti, in cui si registrava un indebitamento dovuto all'aumento delle entrate finali, aumentate di 14 miliardi di euro, e alla riduzione delle spese finali, ridotte di 8,3 miliardi di euro. Il ricorso al mercato finanziario, che è la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti, si attesta a meno 217,6 meno 217,6 miliardi, con un'incidenza sul PIL pari al 12,2 per cento, con un miglioramento di 7,5 miliardi rispetto al 2018. Si conferma quindi il *trend* in calo, registrato già lo scorso anno, di 225,1 miliardi È da evidenziare che sia il saldo netto da finanziare sia il ricorso al mercato registrati dal rendiconto si mantengono entrambi al di sotto del limite massimo fissato dalla legge di bilancio del 2019,

Il dato registrato dal saldo netto da finanziare è da ricondurre a una gestione di competenza che evidenzia un aumento degli accertamenti di entrate finali, con più 14 miliardi di euro rispetto all'anno precedente, dovuto principalmente all'incremento delle entrate tributarie, con un più 12,7 miliardi di euro, e a una riduzione degli impegni delle spese finali pari a 8,3 miliardi di euro. Si conferma altresì la significativa incidenza sul totale degli impegni delle politiche previdenziali, attestatesi al 15,7 per cento della spesa primaria, rispetto al 17 per cento del 2018, e delle politiche economico-finanziarie e di bilancio, che si attestano al 16,1 per cento, di 0,7 punti percentuali rispetto al 15,4 per cento del 2018. L'istruzione scolastica rappresenta il 9,1 per cento della spesa primaria, in leggero aumento rispetto allo scorso esercizio, in cui rappresentava il 9 In percentuale, rispetto agli impegni, si è riscontrato un incremento anche per la missione «diritti sociali», che rappresenta ora il 6,8 per cento della spesa primaria, rispetto al 6,2 del 2018. Nel complesso, si sono registrati accertamenti per entrate finali pari a circa 605,6 miliardi di euro, pari al 103,6 per cento delle previsioni definitive, stimate in 584,78 miliardi di euro. Per quanto concerne la gestione in conto residui, il conto di quelli provenienti dagli esercizi 2018 e precedenti indicava, all'inizio dell'esercizio, residui attivi

Sul versante dei residui attivi rispetto allo *stock* iniziale proveniente dagli esercizi precedenti per 203.940 milioni di euro, sono stati accertati nell'esercizio

In aggiunta a tali residui pregressi, a seguito della gestione di competenza, si sono aggiunti 91.066 milioni di euro di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi, al 31 dicembre, pari a 216.161 milioni di euro, con un aumento di 12.200 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, con un più 6 per cento. Quanto ai residui passivi, sui 140.364 milioni di euro provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati

da pagare. Tali residui pregressi sono aumentati, a seguito della gestione di competenza, per 37.624 milioni di euro, per un totale di residui passivi, a fine esercizio, pari a 114.014 milioni di euro. Nel complesso, il conto dei residui del 2019 espone residui attivi per 216.161 milioni di euro e residui passivi per 114.014 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 102.147 milioni di euro. Sul conto generale del patrimonio (che, come sappiamo, costituisce il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato quale risulta dalla chiusura dell'esercizio), i risultati dell'esercizio evidenziano un'eccedenza passiva di circa 1.916 miliardi di euro, con un peggioramento di circa 13 miliardi di euro rispetto alla situazione patrimoniale del 2018. Tale risultato, pur essendo il più contenuto dell'ultimo decennio, si pone in linea con il *trend* degli ultimi anni, considerato che nel 2018, sul 2017, il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi di euro e nel 2017, sul 2016,

recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020, vorrei sottolineare che, ai sensi dell'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica, il provvedimento in discussione assolve al compito di apportare a metà dell'anno, e quindi nell'esercizio finanziario in corso, l'aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati senza modifiche, ed esaminato dalla 5a Commissione in sede referente e dalle Commissioni competenti per materia in sede consultiva per i relativi pareri, reca l'aggiornamento delle previsioni del bilancio di competenza, formulate ai sensi della legislazione vigente, in relazione, per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime di gettito e, per quanto riguarda le spese, limitatamente alla componente discrezionale in relazione alle esigenze sopravvenute. In sintesi, il disegno di legge in esame, con riferimento alle autorizzazioni al pagamento in termini di cassa, reca l'aggiornamento della consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Le variazioni di bilancio proposte, insieme a quelle apportate fino al 31 maggio in ragione di atti amministrativi,

Le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento sono neutrali ai fini dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, in quanto già scontate nei quadri tendenziali definiti in sede di Documento di economia e finanza 2020. La relazione annessa al disegno di legge evidenzia come, in termini di competenza, le variazioni proposte determinino un peggioramento del saldo netto da finanziare corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta a un valore di meno 302,7 miliardi di euro rispetto a una previsione iniziale di meno 78,6 miliardi di euro. Il peggioramento del saldo netto da finanziare, rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto, per 171,6 miliardi di euro, alle variazioni per atto amministrativo e, per ulteriori 52,5 miliardi di euro, alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento. Nel dettaglio, mi preme sottolineare che il peggioramento determinato dalle variazioni apportate per atti amministrativi è riconducibile agli effetti dei decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento attraverso l'approvazione di apposite risoluzioni relative alle due richieste di scostamento di bilancio presentate dal Governo. Questi determinano nel complesso un incremento delle spese finali per oltre 179,6 miliardi di euro, in parte compensato da un incremento delle entrate finali per circa 8,1 miliardi di euro. Il peggioramento del saldo è dovuto a una proposta di riduzione delle entrate finali per 50,8 miliardi di euro in termini di competenza, riconducibile per quasi 39 miliardi di euro alle entrate tributarie, ed è interamente determinata dal consistente deterioramento della previsione macroeconomica. A tale dato si aggiunge una proposta di aumento delle spese finali per 1,6 miliardi di euro. Sul versante dei residui, il disegno di legge di assestamento provvede ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2019, a seguito della gestione conclusasi nell'esercizio consuntivo. Nel complesso, le previsioni assestate quantificano un aumento di residui finali attivi al 31 dicembre 2019 pari a 216,161 miliardi di euro, a fronte dei 246,389 miliardi di euro di residui inizialmente solo presunti. Per le entrate tributarie, i residui vengono quantificati pari a 108,477 miliardi di euro, con una variazione in diminuzione di 18,667 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali di 127,144 miliardi. Per le entrate extratributarie, i residui ammontano a 106,974 miliardi di euro, con una variazione in diminuzione di 11,538 miliardi di euro rispetto alla previsione iniziale di 118,512 miliardi di euro. Avviandomi alla conclusione, quanto all'ammontare dei residui passivi, quelli riferiti alle spese complessive, comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 752 milioni, sono certificati alla chiusura dell'esercizio 2019 per un importo pari a 114,014 miliardi di euro.

Signor Presidente, mi pare che siamo costretti a parlare di numeri, c'è poco da fare; ma dentro i numeri, che sembrano aridi, c'è tutto: c'è la vita dei cittadini.

- erano rose e fiori; ora invece vedremo dai dati - come si è visto da quanto hanno descritto le relatrici - quanti sono i miliardi dell'assestamento. Il rendiconto si compone della parte bilancio e della parte patrimonio. Il patrimonio dello Stato è negativo per 1.916 miliardi ed è peggiorato di 13 miliardi, ma non mi stupisco: è normale ed è dovuto al debito pubblico. Il rendiconto racconta che c'è stato un accertamento in aumento delle entrate fiscali per 14 miliardi - si parla di accertamento, non è detto che siano stati incassati questo vuol dire aver raschiato il barile, ma ha portato il totale del bilancio, quello che a noi interessa, a 605 miliardi di entrate; poi il bilancio pareggia con l'aggiunta del meccanismo del debito pubblico - scadenze, nuove missioni o rinnovi - a 866 miliardi.

30-40 miliardi erano quelli del *deficit* che era stato approvato nella legge di bilancio, la differenza sono residui), ma già si trattava di 66 miliardi. Il vero problema, nel rendiconto, sono i residui. I residui passivi ammontano a 114 miliardi e questi sono costi, sono debiti; ma, se li abbiamo impegnati per fare investimenti, che vanno fatti

sono in grado di ridurre i residui attivi, che sono una cifra non regolare nel contesto degli importi di bilancio e non è un equilibrio che economicamente possa essere giudicato da un terzo o da un tecnico come un importo esatto.

non si può dire che gli italiani sono ricchi, che ci sono 1.500 miliardi di depositi e 2.500 di ricchezza finanziaria, in obbligazioni e altre forme, perché pensare di toccare questi vuol dire creare

L'operazione Monte dei Paschi, che va in scadenza, genererà una perdita di 10 miliardi; l'INPS è sotto di 26 miliardi; i fornitori non pagati dallo Stato e i debiti non contabilizzati in questo importo sono, a seconda dei diversi sistemi di calcolo, debiti fuori bilancio per 30, 50, 70 miliardi, ma prima o poi anche questi nodi verranno al pettine. Oltretutto, questo meccanismo di non incassare i residui attivi, di dover spendere per i residui passivi e far funzionare la macchina di competenza determina troppa lentezza nel pagare: lo Stato paga lentamente e pagano lentamente tutti gli enti. Questa è la situazione del 2019. Tuttavia, l'assestamento di bilancio, che è un aggiornamento delle previsioni sulla base di cosa è cambiato in base ai dati del rendiconto, raccolta di cifre che a me fanno tremare le gambe: non mi farebbero dormire la notte se fossi il Ministro dell'economia o anche un Sottosegretario (non me ne voglia, signor Sottosegretario). Capiamo tutti insieme - perché il debito non è del Governo e della maggioranza, ma di tutti

L'assestamento prende atto della diminuzione delle entrate finali di 50 miliardi, di cui 39 dalle entrate tributarie, ed è il minimo che si possa dire (credo che sarà anche qualcosa in più).

rinnovi rispetto alle scadenze, che passa da 313 a 563 miliardi di importo totale, con una differenza di 250 miliardi che vanno finanziati. In questo *bailamme* di cifre scompare il saldo primario, che, come sapete, negli anni scorsi era positivo per circa 30 miliardi, ma che poi andava in *deficit* per il pagamento degli interessi di 60-65 miliardi.

ma da quello di cui tratteremo domani apprendiamo che i finanziamenti europei saranno a rate fino al 2026, data dalla quale si comincerà rimborsare; saranno a *tranche,* ammesso che siamo capaci di spenderli. Mi chiedo, quindi, quando e quanto arriverà posto quello che sta succedendo in Europa rispetto all'epidemia: sono prestiti o sono sussidi? Penso - ed è scritto in quello di cui discuteremo domani - che siano tutti prestiti, perché quelli che chiamiamo sussidi saranno la tassa d'iscrizione annua in aumento da parte di tutti gli Stati, per lo meno di quelli che saranno d'accordo. Secondo

Detto questo, faccio gli auguri affinché tutto quello che ho detto nella parte finale del mio intervento non si verifichi, ma si trovi qualche altra soluzione. Nei documenti sinceramente non lo vedo e sottolineo il fatto che tutto quello di cui parliamo a questo riguardo tratta tematiche serie, gravi e importanti che toccano la gente, i primi e gli ultimi. Toccano quindi anche noi, non soltanto la maggioranza e il Governo. Che Dio ci assista!

2020 si svolge quest'anno in uno scenario particolarmente complicato per l'economia e per la società italiana. Questo passaggio è sempre stato molto rituale per la sua tecnicalità. Quest'anno, però, ha una fortissima valenza politica, perché l'impatto del Covid-19 si fa sentire pesantemente nei dati dell'assestamento di bilancio e, di conseguenza, in quello che sarà il bilancio per il 2021. Il rendiconto è uno strumento tecnico per rendere noti al Parlamento i risultati della gestione finanziaria. Costituisce un documento staffetta,

perché costituiscono la base sulla quale poi viene costruito il bilancio per l'anno successivo (in questo caso, per il 2021: verrà presentato nel mese di ottobre o novembre al Parlamento per la discussione).

riassume tutto l'impatto sull'economia della crisi provocata dal Covid e il bilancio che dovremo costruire costruire sarà di svolta e di rilancio, perché partendo da quest'enorme crisi, cercherà di riprogrammare il futuro e la ripartenza dell'Italia. Devo dire quindi che quest'anno più che mai tali numeri assumono un valore politico di speranza e di futuro per il nostro Paese.

la spesa per interessi, che eravamo riusciti a riassorbire dello 0,3 per cento, si assestava al 3,4 per cento del PIL, ma anche il saldo di parte corrente

Tutti questi dati costituivano veramente una base solida sulla quale immaginare una ripartenza per il 2020 e ancora oggi, nonostante lo shock della crisi Covid, sono un punto molto importante per dire che i dati di finanza pubblica in Italia sono stabili. Ciononostante, c'erano delle criticità che si vedevano già nei dati precedenti il rendiconto ed erano rappresentate dalla pressione fiscale e dalle spese. Durante il governo giallo-verde, nonostante la sbandierata *flat tax*, la pressione fiscale è incrementata al 42,4 per cento e ciò ci conferma quanto abbiamo sempre sostenuto, ossia che quella non era una *flat tax* ma niente di più che un allargamento dell'ambito soggettivo del regime forfettario virtuoso introdotto dal governo Renzi. Non molto virtuoso nemmeno l'incremento delle spese in quel periodo, che davano conto di politiche sulle quali abbiamo avuto molto da dire e con le quali non eravamo particolarmente d'accordo. Su queste basi in ogni caso si appoggia il rendiconto dello Stato 2019, che presentava un miglioramento di tutti i saldi sia rispetto alle previsioni definitive sia rispetto ai risultati differenziali: un saldo netto da finanziare migliorato di quasi 23 miliardi di euro rispetto al saldo e di 59 miliardi di euro rispetto alle previsioni definitive; un accreditamento netto, quindi un aumento delle entrate finali, e una riduzione abbastanza significativa delle spese finali; un risparmio pubblico in miglioramento e anche una minore

I dati di questo impatto sono evidenti e negativi. Ciò che mi preme dire è che tutto quello che è stato fatto fino adesso è stato assolutamente indispensabile indispensabile per cercare di tamponare, contenere gli effetti negativi e rilanciare. Tutto questo deve servirci per prepararci a una legge di bilancio che deve essere davvero un provvedimento di svolta, come abbiamo detto

questo non è un momento qualsiasi per quanto riguarda la vita del Parlamento, ma è un momento precipuo, poiché realizza quello specifico adempimento dell'attività del Parlamento che è l'attività di verifica, di controllo e poi, a cascata, anche di indirizzo per il seguito della vita dell'ordinamento italiano. L'adempimento riguardante il rendiconto e l'assestamento è stato rinnovato a seguito della riforma dei documenti contabili e realizzata con la legge n. 163 del 2016. I numeri sono stati elencati e messi in evidenza dai colleghi che hanno parlato prima di me e devo dire con una tecnicalità che è finalmente rispettosa della verità. Sappiamo tutti, chi con più esperienza chi con meno esperienza, che i documenti di bilancio devono rispettare quattro principi fondamentali: la verità, coincidente con la veridicità; il dato della chiarezza; il dato della continuità dei documenti di bilancio; infine, il quarto elemento-principio che è la prudenza. Una discussione sul rendiconto e sull'assestamento deve essere nutrita alla luce di questi quattro principi. I documenti di bilancio che stiamo esaminando risultano veritieri? Risultano capaci di essere nutriti dalla continuità dei dati e delle informazioni? C'è il rispetto del principio della chiarezza? E poi c'è il dato della prudenza? La Corte dei conti in una lettura che sono sicuro fa parte del patrimonio di tutti i senatori ha testimoniato, con il documento cartaceo che abbiamo tra le mani, che questi principi sono stati rispettati. C'è poi un appunto che fa la Corte dei conti rispetto ad un dato riguardante per esempio la materia di competenza della 6a Commissione che presiedo, che sono i cosiddetti crediti-fiscali coincidenti con il cosiddetto magazzino fiscale, di cui anche ieri abbiamo fatto un'operazione verità con il valente e apprezzato nuovo direttore generale dell'Agenzia delle entrate. È emerso come, proprio con il principio della continuità dei documenti di bilancio, quei crediti sono figurativi, nominalistici, non sono in competenza veritieri poiché se messi in esercizio, attraverso l'attività contrattuale con l'Agenzia delle entrate-riscossione, noi correremmo il rischio di avere dei costi effettivi, anziché delle entrate effettive. effettive. Come si coglie allora l'utilizzo di un momento parlamentare sul rendiconto di bilancio dello Stato? assumendo indirizzi e obiettivi nel seguito della vita parlamentare per dotarci di una norma che ci consenta di razionalizzare il magazzino fiscale nella sua parte non veritiera, per fare un'operazione di riordino, altrimenti portiamo avanti una consistenza di potenziale capacità fiscale che non corrisponde alla verità.

14, dispone di un comitato fondamentale che deve essere più oggetto di simpatia sia da parte del Governo che dei parlamentari. Tale articolo pone in campo all'Istat l'esigenza/necessità amministrativa di insediare un comitato che dia luogo a indicatori per la valutazione dello sviluppo equo e sostenibile. I numeri di bilancio cioè, quando vengono declinati con operazioni di spesa, devono dare luogo a valle a indicatori che consentano la misurabilità dello sviluppo equo e sostenibile, anche attraverso una lettura internazionale di pratiche. A tale riguardo dobbiamo fare un'operazione verità. Il documento va approvato poiché è un documento che registra in termini di assoluta eccezionalità una rottura che sul piano planetario viene giudicata come una rottura di civiltà. È chiaro che ciò ha determinato un disallineamento tra le previsioni e l'effettività poi della spesa; evidenza, dal primo collega dell'opposizione al collega che ha parlato prima di me di maggioranza, come alla fine l'operazione finanziaria di risulta sia uno sbilancio circa il coordinamento tra entrate e uscite per circa 300 miliardi di euro. è però il dato aggiuntivo che noi dobbiamo collocare nella nostra riflessione? Dobbiamo porci una domanda: come si ricompone e si ricostituisce il bilancio dello Stato? Noi abbiamo sospeso il bilancio dello Stato per ragioni di necessità. C'è un ammanco dal punto di vista delle entrate perché con voto parlamentare abbiamo determinato una misura di flessibilità sui doveri delle entrate. Abbiamo determinato uno scostamento, che significa indebitamento rispetto al quadro di coordinamento della finanza pubblica italiana ed europea, e anche questo è stato oggetto di voto parlamentare per fare in modo di rincontrare una circostanza di economia reale che restituisca impulso alla produttività, alla ruota dell'economia che deve ricominciare a girare. Che cosa dobbiamo aggiungere, fermo restando l'ordine dei documenti contabili che dobbiamo votare? Noi dobbiamo fare in modo che la spesa della finanza pubblica raggiunga obiettivi in tempi realistici. Questo è il dato. C'era un programma con un nome evocativo nell'ordinamento italiano: Bellezza Italia; non so chi di voi lo ricorda, di sicuro i parlamentari con più lungo corso di me lo ricorderanno. Tale programma riguardava i 6.000 campanili italiani. Sapete dove si trova quel programma? Con tutti i documenti contabili in ordine non ancora genera quell'incontro maestoso di operai, cantieri e cemento, che è la trasformazione della realtà, perché manca un parere di una figura di un Ministero molto esigente, che non voglio citare per evitare qui di creare antipatia e simpatia. È un Ministero che si rifiuta di stare alle regole dei procedimenti procedimenti e che ha in odio i tempi del procedimento amministrativo; li ha proprio in odio, sapendo che la legge n. 241 del 1990 è esattamente trent'anni fa che è stata resa legge dell'ordinamento. A distanza di trent'anni, trenta giorni sono abbondantemente sufficienti per istruire un procedimento e definirlo. Eppure non accade. Questo ci deve portare a fare una riflessione, colleghi adulti *senior* (io mi considero un collega *junior* Casini davanti a me, che quasi mi debilita, giudicando la sua esperienza). Alla luce di questo, vorrei raccogliere l'esperienza di un gigante della contabilità pubblica, Manin Carabba, magistrato autorevole della Corte dei conti, che tante volte ha nutrito i documenti contabili di questo Parlamento. Manin Carabba dice: consideriamo risorsa la risorsa finanziaria, ed è indiscutibile; c'è un'altra risorsa indiscutibile, la risorsa normativa, per la quale noi dobbiamo osare di più. Il provvedimento denominato «semplificazioni» deve essere più esigente nei confronti della semplificazione attesa dal Paese, anche perché la la risorsa normativa non costa: è indeterminata. Soltanto il carico di fatica che impone può produrre una incomprensione. Poi c'è la risorsa organizzativa, la risorsa umana: mancano 500.000 risorse umane alla pubblica amministrazione. Noi non possiamo continuare a produrre programmi, missioni progetti pensando che un commissario *ad acta* risolve tutto; non è così, è un inganno. C'è bisogno di ricostituire una dote di competenze e di allineare modalità procedurali.

Dobbiamo fare in modo che i pronunciamenti dei pareri istruttori vengano trattati come nodi di un procedimento da mettere in priorità in agenda, altrimenti i documenti contabili raccontano di sicuro una verità, ma non è la verità fattuale. Tra i centotrentasei obiettivi misuratori e indicatori che ha vagliato il Ministro dell'economia e delle finanze c'è un obiettivo che parla di impatto reale della spesa pubblica. Noi su quell'indicatore rischiamo di essere un partito unitario di maggioranza univoca, perché non riusciamo a sfondare il niente della realtà dei problemi della cittadinanza. Dobbiamo allora semplificare considerare la modifica di norme pigre e tristi come una grande priorità, per far sì che la spesa pubblica venga rendicontata e giudicata. *(Applausi).* PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

questa è la prima volta che la legge di assestamento e il rendiconto non sono solo un noioso elenco di cifre, ma qualcosa di vivo, perché non è mai accaduto ciò che questa pandemia ci ha messo di fronte. Ripeto, non è mai accaduto, e ci mostra le montagne russe che ha dovuto affrontare l'Italia, come mai aveva fatto prima nel corso della sua storia. Il Covid-19 ci ha gettato nel baratro, ma ha anche fatto emergere la nostra incredibile capacità di recupero e ci ha anche mostrato le qualità di questo Governo. In breve, ecco cos'è accaduto ai nostri conti: un racconto diviso in due, tra ciò che è accaduto prima del coronavirus e quello che è accaduto dopo. Partiamo dal 2019. Per quanto riguarda la spesa per investimenti, il risultato è stato certamente positivo, anche per gli effetti degli interventi di sblocco adottati nei primi mesi dell'azione di Governo. La spesa per investimenti è tornata a crescere dopo quattro anni, segnando un aumento di quasi 3 miliardi di euro rispetto al 2018. Il saldo primario, uno dei nostri fondamentali di cui siamo più orgogliosi in Europa, è risultato positivo ed è pari all'1,7 per cento del PIL (31 miliardi di euro), con una crescita dello 0,2 per cento rispetto al 2018. La spesa per interessi è stata pari al 3,4 per cento del PIL (60,3 miliardi di euro). Il saldo di parte corrente è stato positivo e pari a 27,8 miliardi Se guardiamo ai principali dati aggregati del conto economico della pubblica amministrazione, al miglioramento del saldo concorre principalmente un incremento delle entrate per circa 23 miliardi di euro. del 2019 delle pubbliche amministrazioni sono aumentate del 2,8 per cento; idem per le entrate correnti. In particolare sono aumentate le imposte dirette, in virtù della crescita dell'Irpef, dell'Ires e delle imposte sostitutive, mentre le imposte indirette hanno registrato un aumento per effetto principalmente della crescita del gettito IVA e dell'imposta sul lotto e sulle lotterie. Inoltre, si registra un + 3,2 per cento per i contributi sociali effettivi rispetto al 2018. Il rapporto debito pubblico-PIL è invariato al 134 per cento a fine 2019. La gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2019 un miglioramento di tutti i saldi rispetto alle previsioni definitive, nonché rispetto ai risultati differenziali registrati nel 2018. Il saldo netto da finanziare presentava nel 2019 un valore positivo di circa 2,3 miliardi di euro, con un miglioramento di quasi 22,3 miliardi di euro rispetto all'esercizio 2018. È migliorato il risparmio pubblico e andava bene anche il dato del ricorso al mercato finanziario. Poi è arrivata la pandemia e, assieme ad essa, la catastrofe planetaria dell'economia. Lo *shock* che ci ha investito ha completamente ribaltato lo scenario che inizia a delinearsi dall'inizio del 2020. I dati relativi ai primi mesi dell'anno mostravano, infatti, andamenti pienamente in linea con le migliori previsioni formulate dal Governo e dagli osservatori internazionali. Il *deficit* era al di sotto delle aspettative, il profilo della crescita sulla base di indicatori faceva ritenere che l'economia si fosse stabilmente avviata sul sentiero di una moderata ripresa. Le misure di contenimento dell'epidemia che ci siamo trovati a dover adottare per primi tra le Nazioni europee hanno avuto, purtroppo, un impatto senza precedenti sull'economia: un terremoto potentissimo, amplificato dal fatto che, contemporaneamente, sono state colpite le economie di tutti i Paesi del mondo, non solo dei nostri *partner* europei. Ed è qui che è emerso il Governo. Questa maggioranza ha risposto con interventi tempestivi e di una portata senza precedenti nella storia delle manovre economiche e finanziarie approvate dal Parlamento. Le variazioni di bilancio proposte con il disegno di legge di assestamento, oltre a quelle apportate con atti amministrativi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio, tengono conto degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, ma in modo particolare delle misure straordinarie adottate per contrastare le ricadute negative dell'epidemia. Purtroppo gli effetti sulla nostra finanza pubblica, come fa presente la relazione al disegno di legge di assestamento per il 2020, sono pesanti, con un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni. Si registra nel complesso un incremento delle spese finali per oltre 179 miliardi di euro, in parte compensato da un incremento delle entrate per circa 8 miliardi una riduzione delle entrate finali per 50,8 miliardi di euro. Si sottolinea che tale proposta di riduzione interessa principalmente, per quasi 39 miliardi di euro, le entrate tributarie ed è interamente determinata dal consistente deterioramento delle previsioni macroeconomiche, già illustrato nel Documento di economia e finanza 2020. Ma molti danni sono stati limitati. Probabilmente, l'Italia, per una volta, ha agito meglio rispetto ai suoi *partner* europei e ce lo riconoscono un po' tutti. La Banca d'Italia ha rilevato che, in assenza degli interventi adottati, la contrazione del PIL nel 2020 sarebbe stata superiore di oltre due punti percentuali. Invece, le misure adottate hanno raggiunto larghi strati della popolazione. Una stima piuttosto prudenziale porta a ritenere che siano almeno 1,5 milioni i posti di lavoro salvati finora dalle misure adottate. Al 20 luglio sono state erogate, solo per la parte INPS, prestazioni stimate in 16,5 miliardi di euro in favore di una platea di 12,6 milioni di lavoratori (e io mi sento di essere solidale con il presidente Tridico, un umile professore che sta facendo bene). Le domande pervenute dalle banche al fondo di garanzia sono divenute 918.000 per 61,7 miliardi di euro erogati, di cui circa 784.000 fino a 30.000 euro per 15,5 miliardi di euro. Da una simulazione diffusa dalla BCE nel suo bollettino economico emerge che in Italia, senza gli interventi a sostegno dei lavoratori, la disoccupazione sarebbe balzata al 25

2021-2023 per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione territoriale nel nuovo scenario determinato dal coronavirus. Ci sono misure eccezionali di risposta alla pandemia adottate a livello europeo. Insomma, signor Presidente, la pandemia ci ha cacciati in fondo al *tunnel*, ma oggi ne vediamo, anche se lontana, l'uscita. Questa pandemia è paragonabile è paragonabile all'impatto di una guerra. Per questo nel cercare la ricostruzione di questo Paese dalle macerie economiche e della finanza del neoliberismo c'è bisogno dell'aiuto di tutti,

Colleghi, ricordo che l'assegnazione dei posti alternati ed il distanziamento sono ancora previsti, quindi non vedo perché di colpo ritornino le file piene. Non credo siano previste quattro postazioni in quella sede.

chiusa la votazione.

1.Tab.2.1 propone di spostare risorse dal fondo immigrazione, incrementando quelle destinate agli enti territoriali per interventi di loro competenza. La finalità è quella di dare sostegno agli enti di prossimità, gravemente fiaccati dalla crisi che ha colpito le attività economiche. L'emendamento 1.Tab.2.2 propone di spostare risorse dal fondo immigrazione alla tutela dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. l'intenzione è quella di spostare le risorse stanziate per il *bonus* vacanze, indirizzandole al fondo destinato ai Comuni per il ristoro dell'esenzione TOSAP e COSAP. l'emendamento 1.Tab.2.4 incidiamo sul *bonus* vacanze, ritenendo più opportuno destinare le medesime risorse ai Comuni, per l'esenzione IMU per il settore turismo, misura sicuramente più utile al settore rispetto al *bonus* vacanze. L'emendamento 1.Tab.2.5

Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, i provvedimenti in discussione, sebbene molto tecnici, risultano essere necessari per la vita dei cittadini e la funzionalità della macchina statale.

procedere ad allocare le risorse, in vista del prossimo anno, con la legge di bilancio 2021. Quest'anno la grave crisi legata alla pandemia da Covid-19 ha provocato delle profonde modificazioni nella gestione delle risorse dello Stato. questo passaggio ci permette di costruire un ponte tra la precedente sessione di bilancio, chiudendola, e la nuova sessione di bilancio, riprogrammando le nostre previsioni. Credo che quando il Parlamento è chiamato ad approvare provvedimenti che gestiscono le risorse pubbliche servano la massima serietà e trasparenza. Farlo in un periodo così difficile, inoltre, ci chiama a un impegno ancora più alto e forte. Come dicevo, l'andamento dei conti pubblici ha indubbiamente subito le conseguenze legate alla pandemia. I dati del consuntivo 2019 ci consentivano, infatti, di poter contare su una situazione di stabilità che risultava sicuramente più in linea con le migliori previsioni formulate dal Governo in autunno. Il *deficit* più basso delle aspettative e diversi indicatori economici che riportavano una situazione migliore del previsto lasciavano presagire anche la possibilità di una moderata ripresa. Poi, però, come tutti sappiamo, le misure di contenimento dell'epidemia hanno stravolto completamente quel quadro, ma, nonostante tutto, i numeri dimostrano che l'economia italiana è pienamente sostenibile. E se questo è avvenuto, è stato anche grazie a una serie di interventi che, nel corso degli ultimi anni, hanno permesso allo Stato di tenere sotto controllo la spesa pubblica, efficientandola e recuperando importanti risorse per la collettività, oltre al fatto di poter contare sul sostegno di un'Europa che non ha abbandonato l'Italia e ha garantito la sostenibilità del suo debito pubblico. Tutti noi sappiamo che la situazione che oggi ci viene mostrata dall'assestamento è legata alle condizioni date fino al 31 maggio 2020; fino a quella data si è potuto tener conto anche degli importanti provvedimenti che il Governo e il Parlamento hanno adottato, fatta eccezione per l'ultimo decreto approvato, il decreto agosto. Le variazioni di bilancio che oggi approviamo nella proposta di disegno di legge di assestamento recepiscono infatti anche gli effetti finanziari di tutti quei provvedimenti straordinari adottati per contrastare le ricadute negative dell'epidemia sulla nostra economia (penso ai cosiddetti decreti cura Italia, liquidità e rilancio). Si tratta di interventi che indubbiamente provocano un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta intorno ai 300 miliardi di euro, a fronte dei - 78 miliardi di euro previsti inizialmente. Parliamo di un peggioramento di oltre 224 miliardi di euro del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni, che subisce anche l'influenza di un aumento di spesa, pari a 179 miliardi di euro, legato proprio ai provvedimenti messi in campo finora. Tra questi pesano sicuramente i trasferimenti agli enti pubblici, tra cui 35,4 miliardi agli enti di previdenza maggiori, che sono serviti a coprire gli oneri legati alla cassa integrazione per i lavoratori; senza dimenticare l'importante finanziamento che lo Stato ha garantito alle Regioni e ai Comuni. Per questi ultimi credo che il nostro impegno dovrà continuare con ancora più forza; sindaci e amministratori locali si troveranno a fronteggiare le conseguenze di una crisi economica e sociale che ci obbliga a dare loro maggiori risorse e strumenti per intervenire perché, come sappiamo, sindaci e Comuni sono il *front office* dello Stato rispetto a tutti i cittadini. Come dicevo, approvati questi provvedimenti, il Parlamento potrà entrare in una sessione di bilancio che a mio avviso sarà fondamentale per il futuro di questo Paese. Avremo un compito arduo, ma soprattutto un'enorme responsabilità verso le future generazioni.

Oggi, da quella stessa Europa abbiamo la dimostrazione che l'Italia è e continuerà a essere un punto di riferimento. Con i miliardi del *recovery fund* e con tutti gli strumenti che l'Europa ci ha messo a disposizione dovremo fare la nostra parte: mettere in sicurezza non solo i conti dello Stato ma lo sviluppo, il progresso e il futuro del nostro Paese. Per tutte le ragioni appena esposte, signor Presidente, anche a nome del mio Gruppo Italia Viva-PSI dichiaro il nostro voto favorevole a questo provvedimento.

2019 e l'assestamento di bilancio 2020 rientrano sicuramente tra i temi più importanti che riguardano un'amministrazione, che possa essere quella centrale, come nel caso di oggi, piuttosto che decentrata, come le amministrazioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Si tratta chiaramente di temi che appassionano meno rispetto ai temi politici, nonostante siano questioni comunque molto importanti. Parliamo di documenti tecnici, di numeri, come dicevo prima, dietro i quali il Governo si nasconde per dire che tutto va bene

possiamo certamente dire che, tra i due documenti, c'è uno spartiacque ampio che riguarda la pandemia che stiamo vivendo. Quindi, se i numeri del rendiconto 2019 hanno parametri certamente positivi rispetto a quelli del 2018, i dati dell'assestamento 2020 hanno moltissime negatività, e il peggioramento è dovuto senz'altro al drammatico momento

vera del nostro Paese. Credo che il dato che dovremmo guardare principalmente sia quello relativo al PIL, il nostro Prodotto interno lordo. L'Istat ha dovuto rivedere al ribasso le stime del PIL relativamente al secondo trimestre del 2020, che cala addirittura del 13 per cento rispetto al trimestre precedente per cento rispetto al secondo trimestre del 2019. Confindustria stima che il 2020 si chiuderà con un calo del 9,6 Questo grazie alla ripresa che qualcuno definisce in modo ottimistico di rimbalzo del terzo e del quarto trimestre dell'anno in corso. Una ripresa che sarà sicuramente non omogenea, destinata a lasciare diversi settori indietro: uno per tutti, il turismo che, come tutti sappiamo, rappresenta il 13 per cento del nostro prodotto interno lordo. Sarà comunque questo un percorso di navigazione a vista, dovuto chiaramente anche alla situazione particolare che stiamo vivendo e quindi ai contagi che stanno generando dubbi fortissimi nelle nostre famiglie e nelle nostre imprese, che temono un nuovo *lockdown.*

L'Italia sta vivendo una crisi che è la più importante del Dopoguerra e Fratelli d'Italia sta chiedendo da tempo al Governo un cambio di passo che purtroppo ancora non vediamo. Non possiamo continuare a dilapidare fondi pubblici, risorse, peraltro, come ho detto anche ieri, in *deficit*, né possiamo continuare ad attendere senza far nulla i fondi europei, quei famosi 209 miliardi che ci aspettiamo entro la primavera, forse addirittura entro l'estate prossima. Sono ritardi che potrebbero far comodo ad alcuni partiti della maggioranza, uno per tutti il Partito Democratico, che non vede l'ora di attivare i 37 miliardi del MES, al debito pubblico alle stelle faremo anche 37 miliardi di debito con l'Europa, un grande affare per il nostro Paese. Fratelli d'Italia vi chiede quindi di aprire gli occhi e di fare un rendiconto dei risultati di questo Governo, piuttosto che fare solo i conti riferiti Con un po' di lucidità, vi rendereste conto che continuate a montare e smontare misure promosse dal Governo Conte 1 e a rinnegare quelle promosse dal Governo Conte 2, mi riferisco in particolare alla quota 100 e alle politiche riferite ai decreti sicurezza che, come sappiamo tutti, sono stati smontati nei giorni scorsi. Questo vuol dire chiaramente che non ci sono idee né su come fare la riforma pensionistica, tantomeno su come proteggere i nostri confini e gli italiani da questa immigrazione incontrollata. Si naviga a vista, come dicevo prima, pronti a rinnegare provvedimenti che il partito di maggioranza relativa di questo Parlamento aveva votato convintamente convintamente e non abbiamo ancora capito se vi siete sbagliati o se eravate pienamente consapevoli di ciò che stavate approvando. Su una cosa non si discute più, perché ormai la si dà per scontata, quella misura su cui non si vuole e non si è voluto tornare indietro, che è il simbolo dello spreco per eccellenza, cioè il reddito di cittadinanza, molto caro ai Cinque Stelle. In questi mesi ci siamo sgolati nel dire che questa misura è pensata male ed è finita molto peggio.

I soldi li avete trovati nelle varie leggi di bilancio per finanziare questa misura, ma sinceramente non siamo mai stati e non saremo mai convinti di tutto ciò che avete portato Abbiamo più volte riportato anche in quest'Aula i casi di abuso del reddito di cittadinanza, da parte di gente che non aveva il diritto, o peggio ancora di carcerati, o di chi aveva ville e auto di lusso messe in bella mostra sui *social*, di chi lavorava in nero o di chi spacciava e talvolta anche di chi uccideva. Il rendiconto quindi fatelo a voi stessi, fatelo guardandovi allo specchio, su cosa avete fatto per un'Italia in crisi, che vi chiede riforme strutturali, a partire dal sistema della tassazione fiscale e dalla pesante burocrazia che non siete nemmeno riusciti a risolvere attraverso quest'ultimo decreto approvato e cioè il decreto semplificazioni. Mi taccio sugli investimenti, rispetto ai quali prendiamo atto che il modello Genova è stato un'eccezione e che nonostante i proclami altisonanti nella pratica non si vedono affatto cantieri sbloccati, né tantomeno grandi opere che partono. A tale proposito voglio ricordare gli annunci fatti dal ministro De Micheli, addirittura siamo in attesa di un decreto ministeriale che porti alla nomina di commissari che possano far partire opere che in questo Paese sono ferme da decenni. decenni. Agli esponenti di questo Governo e di questa maggioranza, quindi, diciamo di fare un rendiconto politico. Fatevi un esame di coscienza, dopodiché quando avrete chiara la misura del vostro fallimento, dimettetevi e lasciate la parola agli italiani. Il voto di Fratelli d'Italia sarà contrario sia al rendiconto che all'assestamento. *(Applausi)*.

è un atto di trasparenza molto sottovalutato, anche da noi; invece, come afferma la Corte dei conti, dandone una valutazione assolutamente positiva, è un atto

l'assestamento è uno strumento straordinario perché, mentre negli anni precedenti ci trovavamo di fronte ad aggiustamenti minimali, il Covid fa emergere alcune cose molto significative. Siamo di fronte a un cambiamento radicale, basti pensare alla riduzione pesantissima delle entrate, o al fatto che ricorriamo al mercato per oltre 300 miliardi in più rispetto a quanto previsto e alle spese aggiuntive (mi riferisco alla tabella 1 e alla tabella 5). proposito, vorrei sottolineare che potremmo fare una discussione meno ideologica e meno di posizionamento politico, politico, facendo due esempi molto discussi negli emendamenti e nel dibattito di questi mesi. Se prendiamo la tabella 5 ci accorgiamo

la scelta, l'investimento, la spesa (stiamo parlando di spese) dello Stato e la ricaduta nel territorio.

Bisogna prendere dei progettisti, dobbiamo fare finalmente - anche queste ultime inondazioni ce lo dicono - un piano straordinario, decennale, per la messa in sicurezza del territorio. Ci vogliono i progettisti, le competenze ambientali. Non le abbiamo. Dopodiché non possiamo più permetterci, fra un anno o due, di prendere atto che c'è ancora questo problema.

capace di articolarsi nella rete di decentramento di questo Paese.

d'Europa, l'Italia avrebbe pagato un prezzo più alto dal punto di vista economico. Non è esattamente così e non lo dico per polemica, ma per puntualizzare, perché ci è utile partire da dati della realtà concreta,

non è vero quanto si è sostenuto, anzi, si dimostrerà sempre di più, nei prossimi mesi, che l'azione durissima che abbiamo portato con il *lockdown*, anticipatamente rispetto ad altri Paesi, consentirà - ne sono convinto - una ripresa più rapida. In conclusione, rimane una grande sfida per tutti noi e lo ribadisco ancora. Mi piacerebbe che, al di là delle diverse posizioni politiche, fosse una sfida

È su questo che saremo misurati nei prossimi anni.

Il rendiconto e l'assestamento non rappresentano due atti burocratici, due passaggi tecnici. Sono due pilastri del sistema di bilancio dello Stato, come ha ricordato il collega D'Alfonso dei principi fondamentali della contabilità pubblica. Sono due passaggi fondamentali all'interno dei quali, per quello che riguarda il rendiconto, così come prevede l'articolo 81 della Costituzione, viene data giustamente l'opportunità e la possibilità al Parlamento di verificare se le politiche di bilancio hanno determinato esiti e ricadute economiche e sociali nel nostro Paese. Quindi sono due elementi non tecnici, non burocratici ma di forte valenza politica. Se a questo affianchiamo il fatto che il rendiconto, che consente di portare nell'assestamento i risultati economici, ma anche la base dell'assestamento rappresentano inevitabilmente la base previsionale della legge di bilancio 2021, io credo sia giusto ed opportuno, al di là dei numeri e dei dati che qui sono stati rappresentati dai colleghi che mi hanno preceduto, svolgere alcune considerazioni politiche. Il più importante Il più importante contributo che il Governo ha dato in questo momento - ed è un risultato evidente a tutti - è stato quello di costruire insieme all'Europa un nuovo volto dell'Europa. Dobbiamo ammettere che tanti interventi strutturali e tanti limiti strutturali che abbiamo ereditato dal passato hanno una radice profonda in un'Europa che aveva al centro l'*austerity*, un'Europa che metteva al centro della parola «riforme» tagli, riduzioni di spesa e riduzione di servizi. Questo lo dobbiamo ammettere con grande franchezza tra di noi, invece, attraverso l'azione importante di questo Governo e il cambiamento della dinamica europea, il nuovo volto dell'Europa ci consegni una nuova responsabilità è quella di correggere anche i limiti strutturali che si sono insediati nella pubblica amministrazione. Il collega Errani prima ricordava nelle diverse tabelle un'evidente ricaduta, cioè la difficoltà della pubblica amministrazione di attuare in tempi rapidi le scelte che il Parlamento, anche con la legge di bilancio, individua. Se noi prendiamo i rendiconti, vediamo quanto in molti casi i residui attivi e passivi manifestino una difficoltà di collegamento tra la previsione e l'attuazione. Se poi a questo aggiungiamo anche la valutazione delle ricadute economiche che i ritardi producono o non attuano nel nostro Paese, ci accorgiamo che abbiamo elementi strutturali da risolvere

Questo nella pubblica amministrazione è evidente, perché senza la definizione di una nuova stagione di investimento, anche generazionale, perché le nuove generazioni nella pubblica amministrazione portano con sé innovazione, competenze e nuove tecnologie, non riusciremo a dare velocità alle nostre azioni. Senza dare velocità alle nostre azioni, anche la nuova programmazione europea rischia di non avere tempi utili per la sua attuazione e dunque di non produrre gli effetti positivi ai quali invece noi tutti facciamo riferimento. Dunque credo che il Governo non abbia solo dimostrato di affrontare lo shock più rilevante che questa pandemia ha introdotto; se guardiamo i dati dell'assestamento ci accorgiamo che nessuno di noi avrebbe potuto prevedere ricadute economiche sui saldi di finanza pubblica così violente e così immediate, che di fatto hanno cambiato in pochi mesi la concezione stessa dei saldi di finanza pubblica sui quali avevamo lavorato fin qui. In sostanza, quello shock pandemico, che è diventato uno shock economico-finanziario in tutto il mondo, ci consegna una nuova responsabilità: solo attraverso un nuovo volto dell'Europa riusciremo, con la nuova programmazione europea, ad aprire una stagione nuova. Ecco perché considero questa la più grande opportunità per il futuro. Vi è la prossima legge di bilancio. La Nota di aggiornamento al DEF definisce già l'impianto politico di questa trasformazione. Certo, servono investimenti più importanti nella pubblica amministrazione, perché c'è un ritardo strutturale al quale dobbiamo dare una risposta immediata, perché senza una pubblica amministrazione adeguata e pronta faticheremo a dare attuazione, corpo, velocità e motore ai nostri progetti. Serve una stagione di investimento nella pubblica amministrazione. Credo che questo elemento, unito alla ricerca di un nuovo progetto di sviluppo economico, determini inevitabilmente, con la nuova programmazione, la possibilità di superare i nodi strutturali di questo Paese, anche nelle dinamiche economiche, così da rendere sostenibile l'indebitamento netto che abbiamo costruito. Lo dico ai colleghi senatori: senza queste misure, come già dimostrano i dati di importantissimi istituti economici di valutazione della nostra economia e delle ricadute della pandemia, probabilmente avremmo perso 2 punti in più del PIL. Senza le nostre misure avremmo creato un milione e mezzo in più di disoccupati; senza le nostre misure probabilmente oggi non avremmo nel nostro sistema Paese una capacità di dare resilienza e tenuta al sistema produttivo, industriale ed economico. Senza le nostre misure probabilmente avremmo lasciato al passato una contrapposizione tra lavoro e capitale che oggi è molto meno evidente nel nostro Paese. C'è una consapevolezza in più che lavoro e capitale si tengono, che gli investimenti sulle nuove dinamiche economiche saranno fondamentali per costruire una competitività sui segmenti dell'innovazione, della ricerca, della digitalizzazione, dell'ambiente e della *green economy*. È un pezzo di strada importante. Credo altresì che i 100 miliardi di indebitamento netto, che hanno cambiato i saldi della finanza pubblica in questo Paese, che determineranno nel 2020 una ricaduta che nessuno poteva prevedere prima dello *shock* pandemico, dobbiamo sempre di più affiancarli ad una nuova e straordinaria opportunità che è quella di progettare una nuova dinamica dinamica sociale ed economica nel Paese, finalizzata a costruire competitività e crescita su una nuova concezione di competitività e crescita. Ciò riguarda anche e soprattutto la pubblica amministrazione. soprattutto la pubblica amministrazione. Dobbiamo essere bravi allora ad individuare stazioni appaltanti adeguate, perché non basta dire di assumere, ma dobbiamo sapere dove, come, con quale finalità e con quale obiettivo. ovviamente la stagione per produrre spesa non produttiva, ma la stagione di una spesa produttiva per produrre ricadute economiche concrete che generino occupazione e crescita. Dobbiamo legarla quindi ad obiettivi concreti

nodi strutturali che ci troviamo ad affrontare oggi trovino nel nuovo volto dell'Europa la prima risposta. Credo che lo spazio per chi aveva come avversario l'Europa, per chi immaginava di fare da solo si è azzerato, non c'è terreno di gioco per una competizione interna, per un isolamento del nostro Paese in una condizione di solitudine. Il nuovo volto dell'Europa è la più grande opportunità che abbiamo di fronte per costruire una nuova crescita economica. alla parola riforme oggi dobbiamo dare il significato di un investimento per il futuro delle generazioni, soprattutto per i più giovani, i più giovani, che hanno bisogno di uno Stato che funzioni, di una pubblica amministrazione che abbia al proprio interno generazioni adeguate a poter produrre innovazione, velocità e sviluppo.

per dire che il Governo ha svolto in questa fase pandemica un lavoro prezioso nell'interesse del Paese, ha anticipato misure difficili, si è assunto una grande responsabilità, ma ha anche contribuito a dare all'Europa un nuovo volto e una nuova opportunità per i giovani.

onorevole Vice Ministro, colleghe e colleghi, il rendiconto generale dello Stato è l'atto più giusto e dovrebbe essere anche quello più importante perché ci dice qual è stata la realtà dell'anno precedente e ci permette un giudizio politico su quella che era stata la promessa dell'anno precedente. La promessa si chiama bilancio di previsione, il rendiconto è il mantenimento o meno della promessa, sotto l'aspetto contabile

il raggiungimento dell'obiettivo che si dava la legge n. 196 del 2009, arrivare cioè al giusto equilibrio tra quelle che erano le previsioni di competenza. Dico, anche per i colleghi che non si occupano della materia, che le previsioni di competenza permettevano di scrivere entrate

rapportata comunque alle disponibilità di cassa. Questo è un passaggio verso una modernizzazione del nostro sistema contabile che trova la sua manifestazione anche tramite l'indicazione che ci viene dalla legge n. 196 del 2009, indicando le destinazioni, le responsabilità e quindi la natura delle spese, oltre che delle entrate. Quindi un affiancamento dei due modelli di contabilità. Cosa emerge da questo consuntivo? Emerge un dato di fondo: nel nostro Paese nel 2019 abbiamo avuto il 48,7 per cento del prodotto interno lordo rappresentato dallo Stato. Quindi quasi il 50 per cento della nostra economia è il bilancio allargato dello Stato: questo è un dato molto significativo. Dall'altra parte, c'è una percentuale che ci fa sorridere: 134,8 per cento del rapporto debito-PIL. Discutevamo un anno fa, o anche solo sei mesi or sono, sui decimali di punto;

sui bilanci futuri. Cosa emerge ancora? Ad esempio, emerge un dato per il giudizio politico: maggiori entrate e minore spese, il che contabilmente, dalla lettura di un bilancio, dovrebbe essere un dato molto positivo. Ma diamo anche la lettura politica: queste maggiori entrate quali sono state? Sono probabilmente eccezionali: parlo del condono-rottamazione, certamente. Ma le minori spese, che sono rilevanti (praticamente di 35 miliardi) rapportate agli agli equilibri che avevamo, manifestano purtroppo il grande problema del nostro Paese: l'incapacità di spendere e politicamente l'incapacità del Governo di spendere. Il Governo ha promesso per il 2019 un'azione che - ahimè - non ha mantenuto. Questa è una delle motivazioni del nostro voto contrario rispetto a questo dato. L'altro elemento che possiamo individuare, e che giustamente dovrebbe portarci a fare un'analisi compiuta del sistema, il fatto che il consuntivo ci permette di fare anche un raffronto tra le missioni e le spese; e ci permette altresì, rispetto alle strutture burocratiche che sovente governano più del potere politico, di

di come farla reggere economicamente rispetto agli allievi? È da questo dato che bisogna partire. Dall'altra parte, come possiamo riequilibrare la questione? Si inserisce la questione della scuola pubblica

La situazione di staticità, da un lato, e confusione, dall'altro, la verifichiamo sul passato e - ahimè - sul presente e sui provvedimenti

quando diciamo che alcune cose non funzionano, quando diciamo che il reddito di cittadinanza può essere valso come assistenza ma non è valso come politica attiva del lavoro *(Applausi)*, quando diciamo che le opere pubbliche

ai residui. Infatti, l'assestamento in teoria dovrebbe servire a chiudere i conti dell'anno prima e a portare l'avanzo o il disavanzo al bilancio successivo

miliardi a 216 miliardi: un miglioramento numerico. È un vero miglioramento numerico o è l'incapacità di riscuotere? I residui passivi passano da 140 miliardi a 114 miliardi: vuol dire che lo Stato ha pagato.

perenti. È una situazione che deve essere affrontata alla radice e lo dobbiamo fare proprio perché, rispetto all'assestamento, che in questo caso comincia a incorporare

Veniamo tutti dalla maratona durata più di un mese per il decreto agosto e gli altri provvedimenti e ancora ci aspettano il *recovery*, la legge di delegazione. C'è stato un avanzare

di organizzare e rispettare la tempistica non garantisce un buon lavoro. Questo vale come principio e lo voglio sottolineare. Venendo ai provvedimenti, in merito al rendiconto 2019, ci limitiamo a prendere atto dei risultati conseguiti con riferimento ai saldi di finanza pubblica riferiti all'esercizio 2019, che presentano sia una riduzione del 1,6 per dell'indebitamento netto, ma anche un ulteriore incremento delle spese complessive. Non hanno prodotto alcuna incidenza sul rapporto tra debito pubblico e PIL, che rimane invariato al 134,8 per cento. La pressione fiscale complessiva è al 42,4, ma - come ricordava giustamente il collega Pichetto - comprende anche il discorso della rottamazione. È stata gonfiata, quindi, da un provvedimento che ha avuto

anche in considerazione del fatto che la riforma del fisco è tra le principali politiche di supporto al Piano nazionale di ripresa e resilienza, attualmente all'esame del Parlamento. Riteniamo debba essere oggetto di approfondite e condivise analisi tra le forze politiche

inutile dire quanto questa situazione, soprattutto in questo preciso momento storico, sia insostenibile e metta a rischio la tenuta dell'intero sistema economico nazionale, che si regge appunto sulla micro, piccola e media impresa. Con riferimento all'assestamento di bilancio 2020, non si può evidentemente non segnalare come noi, forze di opposizione, ci siamo sempre dimostrate responsabili nell'affrontare l'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica, offrendo una prospettiva diversa da quelle delle forze di Governo, nel tentativo di arricchire il dibattito sulle misure da adottare, avanzando sempre proposte concrete e fattibili, raccogliendo le istanze del tessuto economico e sociale del Paese, senza la necessità di passerelle mediatiche. Si è poi cercato di agevolare il più possibile - questo dovete riconoscerlo assolutamente - la speditezza dei lavori parlamentari per i procedimenti di conversione dei decreti emergenziali senza meri fini ostruzionistici e con il solo scopo di migliorarne i contenuti, assistendo invece - lo ricordavo ancora ieri durante le dichiarazioni di voto sul decreto agosto - a dei ritardi mostruosi legati alle tensioni interne a una maggioranza sempre più litigiosa e, soprattutto, sorda alle proposte dell'opposizione.

che si sono rese necessarie per affrontare la crisi in atto, votando tre scostamenti di bilancio che hanno prodotto ulteriori 100 miliardi di *deficit* per il solo 2020 e più di 500 miliardi dal 2020 dal 2020 al 2032, portando il rapporto tra debito pubblico e PIL a sfiorare il 160 per cento, tetto che probabilmente sfonderemo con la prossima manovra. Lo abbiamo fatto per senso di responsabilità e perché abbiamo ritenuto indispensabile utilizzare tutti gli strumenti possibili per far fronte alla crisi economica più grave della storia della Repubblica italiana. Abbiamo ritenuto giusto che lo Stato si facesse carico delle difficoltà delle famiglie, dei lavoratori, degli imprenditori e degli enti locali che ogni giorno devono garantire, comunque, i servizi essenziali ai propri cittadini. Non l'abbiamo fatto di certo per vedere le città invase da sfreccianti monopattini - emblema di una maggioranza totalmente sconnessa dalle reali esigenze dei cittadini per consentire mediazioni transattive tra Stato e specifiche Regioni o per favorire l'adozione di micro interventi affatto risolutivi che hanno sostanzialmente dissipato lo sforzo economico che abbiamo chiesto alle prossime generazioni. (*Applausi*). Prima il collega Manca parlava

uno stipendio garantito - parlo della pubblica amministrazione, ma anche di noi - dovrebbero fare propria la frase che pronunciò John Fitzgerald Kennedy: non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo Paese. tutti dovrebbero pensare a essere più seri, a fare di più. Faccio un esempio: in molti uffici della pubblica amministrazione si fa *smart working* e c'è una resistenza a ritornare negli uffici, anche in presenza di tutti i dispositivi e delle garanzie di sicurezza. Ora, io ho raccolto più di una volta testimonianze di cittadini che mi hanno detto di aver bisogno di parlare per risolvere un problema, ma di non riuscire

Ma soprattutto dobbiamo deciderci: semplificare. Non è possibile avere dei residui così importanti e non riuscire a spendere; vuol dire che non siamo efficienti. Bisogna aumentare la produttività e la produttività la si ottiene con i numeri; i premi di produttività vanno dati non perché bisogna darli, ma a fronte di un reale lavoro di efficienza. Questa è la differenza, altrimenti troppe persone pensano di non essere coinvolte nel dibattito e nella ripresa. Resilienza vuol dire essere flessibili e adattarsi,

rischiano in proprio perché rischiano il proprio capitale. Io conosco artigiani che si trovano sull'orlo del fallimento

li pungola comunque a resistere. Perché non esiste questo atteggiamento anche nella pubblica amministrazione? Non si tratta solo dei lavoratori:

esempio degli enti locali - piuttosto che il solito discorso sui forestali. Ci siete, c'è un supporto, c'è un aspetto assistenzialistico, ma il lavoro dovrebbe essere perfetto; i conti dovrebbero essere perfetti; i servizi ai cittadini dovrebbero essere perfetti; i boschi dovrebbero essere puliti; l'assetto idrogeologico anche quello supercontrollato. Invece c'è solamente un approfittarsi, un atteggiamento di menefreghismo che non poteva essere accettato prima e a maggior ragione è inaccettabile in questo momento di crisi dove a tutti viene richiesta

i provvedimenti che oggi siamo chiamati a votare, il rendiconto di gestione per l'anno 2019 e l'assestamento per l'anno 2020, rappresentano il più importante passaggio legislativo per verificare che lo Stato, da un punto di vista gestionale, abbia effettivamente riscosso le entrate previste ed eseguito le spese autorizzate nei termini stabiliti in fase previsionale con la legge di bilancio. un passaggio importante. In termini finanziari viene fissato, approvando il risultato della gestione annuale del bilancio, il flusso della gestione dei conti statali, al fine di consentire il passaggio dalla precedente legge di bilancio a quella successiva; un passaggio a dir poco decisivo - colleghi - viste le sfide imposte dalla pandemia e l'importanza che l'imminente legge di bilancio per il 2021 andrà ad assumere, soprattutto in combinato disposto con il *recovery fund*. Nella composizione dell'imminente manovra, infatti, per continuare a garantire protezione al nostro tessuto economico e produttivo e imprimere una svolta politica di investimenti nel Paese, si profila l'assunzione di impegni di spesa che saranno finanziati dalle risorse del *recovery fund* nel corso del 2021. Il rendiconto di gestione necessità di un'analisi approfondita e di una particolare attenzione, in quanto esprime, attraverso la potenza di numeri, la reale capacità dello Stato di mantenere una sana e proficua interazione con i cittadini, intesi sia come contribuenti sia, soprattutto, come coloro che usufruiranno dei servizi pubblici. Purtroppo, la politica su questo argomento appare da tempo un po' distratta. A volte sembra più facile programmare che entrare nel dettaglio di quello che poi realmente si riesce a concretizzare anno dopo anno. Non ci si chiede mai se le entrate attese siano state riscosse o se le spese autorizzate siano state eseguite. Per non parlare, poi, delle valutazioni che riguardano lo stato patrimoniale del bilancio consuntivo, dove, dal valore dei crediti e da quello dei debiti, si può capire la condizione di salute generale finanziaria dello Stato. Appare pertanto cristallino, cari colleghi, quanto tutto questo sia importante nell'ottica di una tempestiva e proficua spesa delle risorse del *recovery fund*. Non mi stanco mai di sottolineare che il *recovery fund* è un successo enorme ottenuto dal Governo italiano in Europa, con il costante sostegno e stimolo del MoVimento 5 Stelle. Si tratta di ingenti risorse che poggiano su un primo concreto e significativo esempio di solidarietà europea, che si estrinseca nell'emissione di un cospicuo debito comune. Ma proprio per tale ragione, la necessità di una spesa virtuosa di queste risorse è massima. In tale direzione, un esercizio tecnico e apparentemente statico, come l'esame del rendiconto di gestione e dell'assestamento di bilancio, può aiutarci a interpretare e ad affrontare meglio le sfide future lanciate dal *recovery fund* , ormai ribattezzato Next generation EU. Tali considerazioni nascono da una mia precisa volontà di portare all'attenzione di questa Assemblea la necessità di attribuire la medesima importanza al rendiconto di gestione al pari della legge di bilancio. Esiste la malsana abitudine di dare molto più importanza alla programmazione, ma non a questo momento analitico, che è un momento di riscontro di come lo Stato ha funzionato. Ciò potrà accadere solo mediante un cambiamento dell'atteggiamento culturale di tutte le forze politiche qui presenti, affinché possa essere più facile trasmettere le informazioni ai cittadini e renderli pienamente consapevoli di quanto riportato nel rendiconto di gestione. Sono proprio i cittadini che devono capire come abbiamo lavorato, come Stato, lato politico e lato pubblica amministrazione. I valori numerici riportati nel rendiconto sono utili solo nel momento in cui vengono compresi nel loro reale significato. Per esempio, leggiamo che nel 2019 le entrate effettive sono quasi 860 miliardi di euro. Dobbiamo, però, anche tenere conto del valore complessivo dei residui attivi che, al 31 dicembre dell'anno scorso, sono pari a 216 miliardi: euro in più, euro in meno. Ma i cittadini si chiederanno cosa sono i residui attivi. I residui attivi sono entrate previste, accertate ma mai riscosse dallo Stato. Sarebbe giusto capire perché tali somme non sono state riscosse riscosse e cosa si può fare per riscuoterle, visto che sono entrate necessarie per coprire le spese autorizzate dallo Stato nel 2019 e negli anni precedenti. Per meglio capire, voglio fare un altro esempio. Leggiamo che nel 2019 le spese complessive dello Stato ammontano a circa 823 miliardi di euro,

I residui passivi sono voci di spesa autorizzate e impegnate, ma non eseguite. Sarebbe giusto capire perché non sono state spese tali somme e a quali voci corrispondono, visto che sono spese autorizzate dallo Stato nel 2019 e negli anni precedenti e il fatto di non averle sostenute potrebbe avere avuto conseguenze sulla quantità e qualità dei servizi erogati agli stessi cittadini. Se ne deduce - questo passaggio è importante - che i residui attivi e passivi sono parametri che aiutano a comprendere il funzionamento dello Stato nei suoi rapporti con i cittadini. Infatti, l'ammontare complessivo dei residui attivi misura le criticità che lo Stato manifesta nell'incassare le entrate previste, mentre l'ammontare complessivo dei residui passivi misura le criticità che lo Stato manifesta nella capacità di sostenere le spese correnti e quelle in conto capitale, vale a dire gli investimenti dei quali tanto si parla e si parlerà in futuro. Forse ora è più chiaro cosa intendevo dire quando ho parlato dell'importanza del rendiconto di gestione, a maggior ragione in vista dell'imminente legge di bilancio e degli impegni di spesa che verranno presi per i progetti da sostenere con risorse della Next generation L'analisi della gestione di competenza viene completata con due valori apparentemente banali, ma importanti: l'avanzo, che è pari a circa 43 miliardi di euro, e il disavanzo finanziario, pari a circa 103 miliardi. Continuando l'analisi, possiamo leggere i dati dello stato patrimoniale, che presenta un valore attivo complessivo pari a circa 982 miliardi e un valore passivo complessivo pari a circa 2.900 miliardi, con un *deficit* passivo, all'anno scorso, di circa 1.915 miliardi. Anche in questo caso, sarebbe necessario comprendere le cause che hanno generato per lo Stato un così alto ammontare complessivo di crediti e debiti che si sono accumulati nel tempo. Collegato funzionalmente al rendiconto di gestione abbiamo il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato 2020, che serve a definire l'entità effettiva dei residui attivi e passivi che, al momento dell'elaborazione del bilancio di previsione, erano stimabili solo in misura approssimativa. Le variazioni proposte con l'assestamento rivelano un peggioramento del saldo netto da finanziare, pari a circa 302 miliardi di euro, rispetto a una previsione iniziale di meno 78 miliardi. Il peggioramento di oltre 224 miliardi del saldo netto da finanziare è dovuto, per 171 miliardi, alle variazioni apportate per atti amministrativi dovuti agli effetti dei decreti-legge convertiti dal Parlamento, che hanno autorizzato il ricorso all'indebitamento e adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Entrando nel dettaglio, i 171 miliardi - saldo netto da finanziare, come ho detto prima - derivano da un incremento delle spese, pari a circa 180 miliardi, e a maggiori entrate per 8 miliardi. Al peggioramento del saldo netto da finanziare contribuiscono anche le variazioni proposte dal presente disegno di legge di assestamento per 52 miliardi, dovute principalmente a una riduzione delle entrate finali per oltre 51 miliardi. Queste variazioni tengono conto del nuovo quadro macroeconomico definito nel Documento di economia e finanza di aprile 2020, che indica un peggioramento delle condizioni economiche dello Stato conseguente alle misure di contenimento adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. I numeri che finora ho portato alla vostra attenzione hanno un forte valore informativo, in quanto evidenziano un quadro economico, finanziario e patrimoniale con delle criticità che vengono da lontano, ma aggravate dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Tali valori sono stati recepiti dal Governo, che sta già lavorando per realizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, utilizzando le risorse che saranno messe a disposizione dall'Unione europea con il *recovery fund*. Uno degli elementi portanti dell'azione del Governo riguarderà specificamente il rapporto Stato-cittadini, che dovrà migliorare attraverso l'efficientamento della pubblica amministrazione, con l'adozione di un moderno modello gestionale. L'aspetto della formazione dei dipendenti è fondamentale, come lo è anche l'assunzione di figure tecniche e non più In tal modo, sarà possibile avere un'organizzazione pubblica centrale e locale più performante ed efficiente capace di soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini, facendo fronte alle loro esigenze e all'evoluzione delle stesse, contenendo al contempo la spesa pubblica, rendendola funzionale al modello adottato, che potrà essere misurato nel tempo dalla riduzione complessiva dei valori residui attivi e passivi riportati nei futuri rendiconti di gestione. Il concetto di spesa funzionale - sottolineo questa voce - dovrà prendere il posto di quello dei tagli lineari che si sono dimostrati inefficaci e pericolosi per lo Stato sociale. Si sta altresì lavorando per potenziare la digitalizzazione della pubblica amministrazione, sia nei processi interni sia nei rapporti con i cittadini, favorendo l'interazione tra le banche dati pubbliche. Ciò determinerà una maggiore efficienza, e quindi minore spesa pubblica, e una maggiore velocità nell'erogazione dei servizi da parte dello Stato. Un altro intervento al quale il Governo sta lavorando è la riforma fiscale, necessaria a superare il rapporto conflittuale con lo Stato, dovuto a un sistema fiscale datato, inadeguato a rispondere a esigenze di riscossione efficace dei tributi che dovrà tenere conto anche dei cambiamenti avvenuti nel sistema economico e finanziario nazionale e mondiale degli ultimi decenni; una vera e propria rappacificazione graduale e continua che passerà attraverso provvedimenti legislativi tesi a rivedere le logiche del fisco in ottica sempre meno vessatoria e che avrà come effetto anche la riduzione del fenomeno dell'evasione fiscale. Il Governo e il Parlamento stanno lavorando per rafforzare e rilanciare in tempi brevi il Paese, attuando le misure e le riforme che da tempo si attendevano e che in modo incomprensibile negli ultimi decenni sono state disattese. Abbiamo l'occasione irripetibile di rendere l'Italia un Paese moderno ed evoluto, in grado di garantire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini su tutto il territorio, di ridurre il divario economico, sociale e infrastrutturale tra Nord e Sud, di trattenere i nostri giovani e di attrarre investimenti stranieri. Non possiamo permetterci di sbagliare e di perdere altro tempo. Lo dobbiamo ora a noi stessi e alle future generazioni. Dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a entrambi i provvedimenti

La seduta è ripresa. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 15 ottobre. Nella seduta di oggi avrà inizio la discussione generale della legge di delegazione europea 2019 e e delle connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La giornata di domani sarà dedicata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo alle Commissioni bilancio e politiche dell'Unione europea, chiamate ad esaminare le linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza. La discussione della relazione sul predetto documento, per la quale sono state ripartite sette ore, comprensive delle dichiarazioni di voto, avrà luogo martedì 13 a partire dalle ore 9,30. Le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2020, già previste per le ore 15,30 di martedì, avranno luogo a partire dalle ore 17. Per la replica del Presidente del Consiglio, orientativamente intorno alle ore 19, e per le dichiarazioni di voto è prevista la trasmissione in diretta televisiva. Il calendario dei lavori della prossima settimana prevede inoltre il seguito della discussione della legge di delegazione europea 2019 e delle connesse relazioni, nonché l'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020

abbiamo messo in evidenza più volte la totale assenza di programmazione da parte del Ministro su questo tema, che era naturalmente fondamentale.

le scuole sono ripartite, ma in molti casi mancano gli insegnanti, mancano le aule con gli spazi adeguati e in tantissimi casi mancano i famosi banchi promessi (solo il 12-13 per cento sono stati ad oggi consegnati). In molti casi il programma scolastico non è ancora cominciato, tenendo presente che a marzo, soprattutto sul tema degli insegnanti, la Lega aveva presentato un programma chiaro che avrebbe consentito, se attuato in tempi rapidi e certi, che l'anno scolastico potesse partire con tutti gli insegnanti. Purtroppo, Presidente, quando si agitano è perché hai messo il dito nella piaga. Di conseguenza capisco che l'agitazione sia molta. Continuate pure ad andare avanti che ci fate un favore. Soprattutto non si può pensare di colmare gli spazi della mancanza di ruoli attraverso i concorsi, perché sappiamo che hanno tempi lunghissimi. C'era una grandissima occasione per poter stabilizzare gli attuali Questo è quello che noi chiediamo, così anziché mormorare dietro il microfono, avranno la possibilità di intervenire per sostenere che non hanno Seconda richiesta che facciamo: durante la Conferenza dei Capigruppo c'è stata la disponibilità da parte del Ministro e della maggioranza a voler comunque accontentare la nostra richiesta, ma in un tempo troppo lungo a nostro giudizio.

dove ci sono stati lanci di materassi e sono stati dati alle fiamme diversi oggetti - la polizia non riesce più a contenere quelle persone - ma soprattutto

e solo negli ultimi giorni un medico si è accorto che l'immigrato non stava bene. Questo lo diciamo con estrema chiarezza, perché di tutto è stato detto in quest'Aula e non solo nei confronti della Lega e di Matteo Salvini, ma quando gli immigrati erano sulle navi, per cui avete mandato a processo Matteo Salvini, donne, bambini e persone malate venivano fatti subito sbarcare e assistiti. Questo è quello che faceva il disumano, il cattivo, il razzista, quello che va processato. Questo è quello che facevamo noi: assistenza alle persone malate. Invece con gli accoglienti e benpensanti del Governo giallo-rosso

Bene: se questi sono i risultati, il ministro Lamorgese venga subito a riferire dello scandalo e della vergogna cui abbiamo assistito in questi giorni.

*(PD)*. Signor Presidente, capisco ora l'atteggiamento tenuto anche in Conferenza dei Capigruppo. In effetti è comprensibile che i risultati delle recenti elezioni abbiano creato una che si traduce in un intervento sgangherato completamente fuori tema, ma che ha così voluto provocare confusione all'interno dell'Assemblea. In realtà parto dalla seconda richiesta rivolta al ministro Lamorgese, che ha immediatamente dato disponibilità a venire a riferire in Aula. L'abbiamo chiamata oggi, non è stata avvertita e la settimana successiva sarà qui a riferire perché noi stessi abbiamo a cuore la comprensione degli eventi recenti rispetto alla situazione che si è creata, nello specifico su quella nave, così come vorremmo un aggiornamento sulla situazione relativa alla vicenda dell'immigrazione e anche sulle questioni riguardanti i rapporti con l'Europa, compresi i risultati che stiamo ottenendo con questo Governo sulle ricollocazioni di tutti gli sbarcati. Credo che, se siamo minimamente seri, siamo ovviamente disponibili ed, anzi, io credo si debba ringraziare

Commenti).* Apprezzo l'applauso del senatore Romeo perché so che condivide tali questioni. Allora prima di parlare in Assemblea, si deve fare mente locale. La sfiducia è una cosa importante. Credo che la scuola stia partendo

mentre sono una cosa molto seria, la Lega ne ha presentata un'altra sul ministro Gualtieri che, siccome ora non è più di moda, non gli interessa calendarizzare. Prendiamo atto di questo atteggiamento, lo giudichiamo per quello che è, strumentale, dopodiché in Aula affronteremo i temi con la nostra costante sobrietà. *(Applausi)*. Signor Presidente, «L'illeggibilità della firma depone per la presenza di sensi d'inferiorità vissuti nel passato e non ancora del tutto risolti». Questa è un'indagine grafologica sulla firma del ministro Azzolina, che è solo la punta dell'*iceberg* di un'oscena campagna denigratoria

il "ballario" di cui ho sempre parlato; anzi, dov'è chi utilizza sempre questo "ballario"? L'avete lasciato a casa e non sta parlando qui. C'è la fornitura di 11 milioni di maschere al giorno; c'è la fornitura di gel

detto: «I miei figli. I miei figli»? Vi dovreste vergognare, dunque, di non partecipare a questo clima costruttivo e di seminare odio e discredito rispetto a una persona che sta facendo del suo meglio, attaccata da tutti, dai sindacati, dai partiti politici, dalle persone. È una cosa vergognosa. Signor Presidente, al di là dei temi, quello che sta subendo il ministro Azzolina è un attacco vergognoso, senza precedenti. *(Applausi)*. Sfido ad avere contezza e a produrre testi riguardo all'amministrazione della scuola, che

dare fastidio che si recepiscano le indicazioni del Presidente della Repubblica. Su questo argomento *(Commenti)* dobbiamo ragionare insieme, perché i morti i morti sono morti; vanno fatte indagini, vanno accertate le responsabilità e verranno a riferire tutti i Ministri del caso: nessuno deve speculare su questo. Tuttavia, per quanto riguarda la legislazione - e questo è il nostro compito - vigono ancora quelle norme. Se è da cambiare qualcosa, si cambierà. Dovreste collaborare anche su questo, senza utilizzare campagne - come dicevo denigratorie, cercando del facile consenso su questi argomenti. Lo vuole il Paese, non lo vogliamo noi e lo sapete benissimo. Far mancare il numero legale rispetto alla proroga del decreto emergenza è un fatto che capite solo voi. Fuori da qui la gente vuole essere tranquilla, sicura e non vuole che si utilizzino degli espedienti della vecchia politica per mettere in difficoltà una maggioranza che sta portando avanti il Paese senza la vostra collaborazione. *(Applausi. Commenti)*. Ma tanto, con voi o senza di voi, andremo avanti.

riepilogo. Senatore Romeo, lei chiede di inserire, oltre a quanto da me letto dell'attuale calendario, la discussione sulla mozione di sfiducia al ministro dell'istruzione Azzolina e sulla mozione di sfiducia al ministro dell'interno Lamorgese.

Presidente, signor Ministro, onorevoli Sottosegretari e colleghi, portiamo in Assemblea oggi un importante provvedimento legislativo, che rappresenta uno dei cardini nel rapporto tra le istituzioni italiane e le istituzioni europee. La legge di delegazione europea, che consente il recepimento di 38 direttive e l'adeguamento a 17 regolamenti dell'Unione europea, ha comportato un lavoro robusto, meticoloso, attento all'ascolto di oltre 90 interlocutori, nonostante le condizioni particolari dovute alla pandemia. Di questo lavoro poderoso desidero ringraziare il ministro Amendola e il sottosegretario Agea, che ci ha accompagnato passo dopo passo; il presidente Licheri, il vice presidente Bossi e tutti i membri della Commissione politiche dell'Unione europea, di maggioranza e opposizione; la relatrice Gaudiano, che ha curato le relazioni programmatiche e consuntiva in modo sintonico con la legge di delegazione. Ringrazio il neo presidente Stefano, sotto la cui Presidenza abbiamo percorso l'ultimo miglio. Sono grato poi al segretario della Commissione e a tutto il suo *staff*, che ci hanno affiancato con professionalità e impegno. Ringrazio tutti per la coralità. Sono davvero fiero e felice di essere uno degli attori di questo passaggio legislativo. Il disegno di legge in esame è particolarmente importante per due ordini di motivi. Innanzitutto, consente all'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, rispondendo all'obbligo di dare attuazione alle direttive e ai regolamenti, riducendo così il numero delle procedure di infrazione nei confronti dell'Italia ed evitando l'apertura di nuovo contenzioso. Il provvedimento è importante anche dal punto di vista del merito, perché ci sono direttive che nella loro attuazione vengono modificate e introdotte perché si tratta di ambiti che interessano direttamente la vita dei cittadini italiani e delle imprese. Le direttive da recepire riguardano, infatti, servizi *media* e audiovisivi; il diritto d'autore per le pubblicazioni *online;* l'uso delle fonti energetiche rinnovabili; il ricorso all'autoproduzione elettrica; la concorrenza del mercato interno anche tra imprese agricole; i requisiti prudenziali richiesti alle banche e ai fondi di investimento; il benessere degli animali; la tutela dell'ambiente; la vigilanza sui dispositivi medici; la cybersicurezza; il prodotto pensionistico europeo; l'insolvenza degli individui; le condizioni di lavoro e l'equilibrio con la vita familiare; la gente di mare; le infrastrutture stradali e altro. Conseguentemente, il lavoro della 14a Commissione si è svolto - lo voglio ribadire - con la massima apertura nei confronti del contributo costruttivo da parte di tutti i senatori appartenenti a tutte le forze politiche per portare avanti un lavoro corale e condiviso che sia a beneficio dell'Italia e dei cittadini italiani. La Commissione ha integrato e migliorato il testo del provvedimento approvando 113 emendamenti e accogliendo 54 ordini del giorno. Circa la metà degli ordini del giorno (29) riguarda l'articolo 9, relativo all'attuazione della cosiddetta direttiva *copyright*, su cui si è ritenuto di non adottare modifiche al testo. I restanti ordini del giorno riguardano l'attuazione del codice delle comunicazioni, la direttiva sulle fonti rinnovabili, la direttiva sulle plastiche monouso e altri argomenti specifici. Vorrei evitare un esame articolo per articolo e darei per letti i vari articoli,

Penso siano stati oggetto di emendamenti in Commissione e poi in Assemblea. Quindi, vorrei evitare di esaminare articolo per articolo

Il mio auspicio e il mio invito sono, dunque, a procedere, anche in quest'Assemblea, a sostenere nel modo più ampio e con il contributo più largo di tutti i Gruppi e dei singoli senatori l'approvazione della legge di delegazione. Signor Presidente, senatori, Governo, congiuntamente al disegno di legge di delegazione europea il Regolamento del Senato prevede che siano esaminate anche le relazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Abbiamo quindi al nostro esame la relazione consuntiva per il 2019 e la relazione programmatica per il 2020, su cui la 14a Commissione mi ha conferito il mandato a riferire a questa Assemblea

poiché riflette la visione generale del Governo sulle prospettive future dell'Unione europea e indica le sue intenzioni politiche sui singoli *dossier* europei. Entrambe le relazioni trattano dell'intero panorama delle politiche dell'Unione europea, alle quali l'Italia partecipa attivamente e dalle quali discendono obblighi giuridici da adempiere e indirizzi comuni europei a cui informare le nostre politiche nazionali interne. Mi limito in questa sede a soffermarmi su un aspetto che ritengo di fondamentale importanza e che non sarà mai evidenziato a sufficienza, ovvero l'esigenza di dedicarsi in modo primario alla fase ascendente di formazione e di negoziato della delegazione europea, che precede la definitiva adozione ed entrata in vigore in conseguenza della natura vincolante dell'obbligo giuridico di dare attuazione alla legislazione (regolamenti e direttive) che viene adottata dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo, peraltro con la partecipazione attiva dei nostri rappresentanti in seno alle istituzioni europee. Ritengo che una più ingente e incisiva quantità di risorse, di tempo e di energie debba essere dedicata a questa fase sia da parte delle strutture del Governo, che già fanno molto, ma che debbono ulteriormente potenziare questo impegno per porsi alla pari dei principali attori statali nell'Unione, sia da parte del parlamentare. Con riguardo alla parte parlamentare mi riferisco anche ai nostri colleghi eletti al Parlamento europeo, con i quali dovremmo dialogare con cadenza regolare, in modo sistematico e approfondito, creando sinergie di collaborazione e sostegno reciproco; un dialogo in cui noi potremmo dare un apporto dalle istanze nazionali e regionali, di cui siamo rappresentanti, e in cui potremmo al contempo ricevere dai deputati italiani elementi informativi preziosi, punti di vista e opinioni in grado di arricchire la nostra capacità di esame in fase ascendente delle proposte legislative legislative europee. È un ruolo, quello dei Parlamenti nazionali, al quale i trattati europei attribuiscono un valore importante, e non solo per l'effettivo intervento consultivo nel processo legislativo europeo, ma anche per l'importante valenza di stimolo e indirizzo al Governo e per il ruolo di coinvolgimento e avvicinamento delle politiche europee ai cittadini e al territorio nazionale e regionale; un ruolo tanto più importante quanto più risulta evidente la problematicità, soprattutto a livello livello regionale e locale, nel dare corretta attuazione alla normativa europea. L'Italia infatti risulta agli ultimi posti nella classifica delle procedure di infrazione, non tanto per mancata o ritardata attuazione delle direttive, ma per successiva violazione delle stesse. In buona parte si tratta di infrazioni in cui la responsabilità risiede a livello regionale o locale. All'ultimo aggiornamento del 2 luglio 2020 il totale delle procedure aperte ammonta a 91, di cui ben 69 sono quelle derivanti dalla violazione del diritto europeo, mentre solo 22 sono quelle per mancata attuazione. È evidente, quindi, che l'Italia ha un problema di adattamento alla normativa europea, il cui miglioramento potrebbe molto giovarsi di una maggiore dedizione alla fase ascendente. Le procedure di infrazione rappresentano un problema che, oltre ai risvolti giuridici, ha anche degli importanti risvolti economici, se si considerano le sanzioni che l'Italia sta già pagando e che rischiano di aumentare, con le possibili ulteriori sentenze di condanna, che si prospettano. Pendono infatti sull'Italia tre procedure di infrazione *ex* articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancata attuazione di una precedente sentenza di condanna della Corte di giustizia, che sono appunto quelle suscettibili di infliggere al nostro Paese sanzioni pecuniarie. Quando queste tre giungeranno a sentenza, si aggiungeranno alle sei sentenze già emesse, per le quali l'Italia sta già pagando le relative sanzioni pecuniarie, che ammontano a circa 150 Si tratta delle sentenze in materia di contratti di formazione e lavoro, discariche abusive, rifiuti in Campania, acque reflue urbane, mancato recupero di aiuti di Stato per Venezia e Chioggia e mancato recupero degli aiuti di Stato connessi agli alberghi della Regione Sardegna. Le tre procedure pendenti, invece, riguardano il mancato recupero di aiuti di Stato e il trattamento delle acque reflue urbane. Il testo della relazione consuntiva relativa all'anno 2019 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti. La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali. La seconda parte del documento, quella più consistente, è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali. La parte terza, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2019 e dello stato di attuazione del ciclo settennale 2014-2020. La quarta parte è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea, nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento. Infine, la relazione consuntiva è completata da cinque allegati, di cui il quarto contiene l'elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera dei deputati, in fase ascendente, sulle proposte legislative dell'Unione europea. La relazione programmatica per il 2020 è stata presentata alle Camere il 24 gennaio 2020, in un contesto pre-Covid e appare pertanto evidentemente superata dal mutato quadro programmatico europeo e nazionale, a fronte della situazione di crisi economica e sociale derivante dalla pandemia del coronavirus. una situazione programmatica, che è inoltre in continua evoluzione, in base all'evoluzione della pandemia e in base ai negoziati in corso sui diversi strumenti normativi e finanziari, messi in atto dalle istituzioni europee in risposta alla crisi. Appare pertanto opportuno prendere atto del quadro programmatico delineato che riprendeva le principali sfide che la nuova Commissione europea aveva voluto assumere in via prioritaria, ovvero l'obiettivo di recuperare competitività globale, da raggiungere attraverso due direttrici fondamentali: la trasformazione industriale del *green deal* europeo europeo e la sinergia tra le imprese europee per lo sviluppo, in grado di contrastare la competizione spesso sleale degli altri grandi attori globali. Il testo della relazione è preceduto da una sintesi in cui si evidenziano le singole posizioni e azioni che il Governo intendeva portare

alle priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. La terza parte è rivolta al tema della dimensione esterna dell'Unione e illustra quindi gli orientamenti governativi in materia di politica estera e di sicurezza, nonché in materia di allargamento, politica politica di vicinato e collaborazione con i Paesi terzi. La quarta parte è dedicata alle strategie di comunicazione e di formazione del Governo, in merito alle attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea. Infine, la quinta parte è dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee dal Comitato interministeriale per gli affari europei e al tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea con la consueta finestra sulle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione. Completano il testo due appendici in cui si riportano il programma

Avverto che le proposte di risoluzione alle relazioni programmatica e consuntiva potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

prodotte, distribuite e consumate, mentre emergono costantemente nuovi modelli di *business* e nuovi attori. Inoltre, sappiamo che la rete e il digitale rappresentano straordinari strumenti di diffusione di contenuti, conoscenza, relazioni

riferisco al non riconoscimento del valore delle produzioni intellettuali, che invece sono un punto fondamentale per la nostra economia e la nostra convivenza democratica.

Basta guardare agli ultimi mesi e a quanto il digitale sia stato centrale per garantire, almeno in parte e con tutti i limiti che abbiamo sperimentato, la continuità scolastica, il lavoro, i consumi, l'informazione e lo stesso bisogno esistenziale per la nostra socialità. Certo, ci siamo anche accorti di quanto lo spazio digitale non sia accessibile a tutti nello stesso modo e di come non tutti e non tutte siano nelle condizioni di beneficiarne equamente. è una delle ragioni per le quali, già nei mesi scorsi, nel pieno dell'emergenza Covid-19, abbiamo spinto con forza per arrivare il prima possibile - al massimo entro questo autunno - a recepire la direttiva europea sul *copyright,* che, oltre a essere una scelta di civiltà mirata a garantire la qualità, l'equità e la sostenibilità democratica dell'innovazione digitale, è anche una risposta concreta alle enormi difficoltà che il coronavirus ha creato e sta creando al mondo della cultura e dell'informazione. Con questa direttiva, per la prima volta l'Europa ha riconosciuto l'intreccio fondamentale tra il diritto degli utenti ad accedere alle opere in Rete, al fine di citazione, critica, rassegna, e quello degli autori e delle autrici a ottenerne il giusto e sacrosanto riconoscimento economico da parte delle piattaforme *online*. *(Applausi).* Come sapete, i cosiddetti giganti del *web* li utilizzano e, attraverso la pubblicità, ottengono notevoli guadagni. Si è lavorato alla ricerca di un giusto equilibrio tra interessi diversi di tutti i soggetti coinvolti, tenendo insieme il diritto al libero accesso alla Rete e alle nuove tecnologie con la tutela della produzione intellettuale: un lavoro confluito nella direttiva approvata dal Parlamento europeo nel marzo 2019, confermata dal Consiglio della UE che oggi ci apprestiamo anche noi a recepire

democrazia dignità delle persone e del lavoro, che sono i fondamenti delle nostre istituzioni europee e nazionali. Una vittoria dell'Europa che crede e sostiene la creatività, la cultura, l'arte, la libera informazione, ma è anche una vittoria dei cittadini e delle cittadine che possono usufruire gratuitamente dei contenuti che vengono pubblicati in Rete. La direttiva, infatti, prevede, qualora detti contenuti comportino degli introiti - sono le piattaforme, escluse quelle di nuova costituzione (pensiamo alle *startup*, ai blog, agli *account* personali) ed enciclopedie *online* senza scopi commerciali come Wikipedia di doverli corrispondere a chi ne detiene la proprietà intellettuale: agli artisti, ai giornalisti, agli scrittori, agli sceneggiatori, agli editori. Insomma, la legge di delegazione europea di cui avviamo la discussione oggi è quindi davvero coerente rispetto all'obiettivo generale che la nostra legislazione ha per potersi progressivamente adeguare a questo nuovo contesto. Considero questo un punto politico importante. Tutto ciò senza limitare o ostacolare l'evoluzione tecnologica - anche questo è un punto importante né compromettere la libera circolazione delle idee, che è un caposaldo non solo della Rete, ma della nostra stessa Costituzione; ma insieme, tenendo davvero questo intreccio, difendendo il patrimonio di conoscenza generato da artisti, giornalisti, traduttori, autori in genere. La legge sul *copyright*, insomma, è una forma virtuosa ed equilibrata di regolamentazione; non comporta alcuna limitazione alle potenzialità offerte dal *web*, anzi, aumenta piuttosto la pluralità dell'offerta. Tutelare chi produce contenuti culturali, editoriali e artistici significa, infatti, investire nella produzione culturale, editoriale e artistica, favorire la pluralità dei contenuti stessi, la sostenibilità economica del lavoro intellettuale e la trasparenza della concorrenza in ambito digitale, punto politico della modernità. È quindi una legge importante, una legge di civiltà, come dicevo, che pone fine a una confusione in cui ad avvantaggiarsi sono stati finora solo alcune grandissime aziende del *web*, a discapito di tutte quelle realtà editoriali, culturali e artistiche escluse dalla fruizione del ritorno economico del prodotto del proprio capitale umano, e che da oggi potranno invece vedersi riconosciuto un giusto compenso, dignità sociale, lavorativa e personale. questo serve alla qualità culturale del nostro Paese, di cui, tra l'altro, il nostro Paese è autenticamente invidiato in Europa e nel mondo. *(Applausi).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, ringrazio anch'io per il lavoro che è stato fatto nella Commissione politiche dell'Unione non faccio parte, ma ho seguito la vicenda del diritto d'autore che, con l'articolo 9, è uno dei punti importanti di questo disegno di legge di delegazione europea. Ringrazio i relatori, il senatore Pittella in particolare, con il quale abbiamo avuto modo di approfondire in corso d'opera la vicenda. È una questione importante, che parte da una dura battaglia perché, colleghi, voglio che restino agli atti anche le responsabilità dei giganti del *web*, che stanno facendo un'azione di *lobbying* asfissiante in tutto il mondo, in tutto il Pianeta. Abbiamo una morsa: da una parte, la Cina con la via della seta e con tutti i pericoli anche sanitari, la sua voglia di egemonia e di colonizzazione che si estende fino al tentativo di acquisto dei porti italiani; dall'altra, i giganti del *web* esentasse che, da Occidente, marciano tritando tutto e tutti senza pagare tasse. Questa è la realtà. E saccheggiano saccheggiano la creatività, saccheggiano il prodotto intellettuale, mettono in ginocchio il mondo editoriale, saccheggiano la produzione degli artisti, del cinema, dei musicisti; mondi che, peraltro, in questa fase stanno già vivendo una difficoltà enorme, perché tutte le attività artistiche, le attività pubbliche, le sale cinematografiche, le produzioni che le alimentano soffrono per la

poi vuol dire diritti d'autore, incassi, denaro per tutti gli ambiti della creatività. La direttiva sul diritto d'autore è stata molto contrastata. A un certo punto qualche anno fa, quando la si discuteva a Bruxelles, non si trovavano avvocati liberi perché le *lobby* dei grandi giganti della rete avevano ingaggiato tutti gli avvocati di Bruxelles, tutti i consulenti per impedire che chi si difendeva dall'altro lato (autori, editori, musicisti) trovasse, nello scontro da un lato una *lobby* potente e dall'altro la creatività, delle persone a cui affidarsi. C'è stato uno strapotere di Amazon, di Google, di Facebook, di tutta questa gente che non paga tasse ed è una vergogna che in Italia e in Europa si continui ad applicare la *web tax*. I signori di Amazon, a fronte di un fatturato in Italia di 4,5 miliardi di euro, di euro, hanno pagato l'anno scorso 11 milioni di euro di tasse, lo 0,2 per cento. Io accetterei di pagare il 20 o il 30 per cento di tasse, visto che ne pago di più, giustamente, in percentuale sul mio reddito.

che paghino il diritto d'autore. E se prendono articoli di giornale che gli editori fanno scrivere a giornalisti inviati in Afghanistan, in America, a Singapore, a Hong Kong a raccontare una cronaca, a testimoniare i fatti della storia, che costano (il giornalista va, racconta, rischia) non è possibile che quel contenuto poi lo si possa ritrovare in Rete. È bellissimo,

Bisogna tutelare il diritto d'autore, che è questo, perché senza la creatività la vita dei popoli diventa più arida. Anni fa Celentano, che ogni tanto riscopre questo problema quando tocca anche i suoi interessi, scrisse un bell'articolo sul «Corriere della Sera» e disse - la citazione può sembrare impropria, ma parliamo di autori - che se il pane non si pagasse non ci sarebbero i fornai. Se si potesse andare a prendere al banco del pane il pane gratis, chi lo dovrebbe fare questo pane? Chi dovrebbe raccogliere il grano, macinarlo e lavorare di notte? Nessuno farebbe il pane se il pane non si pagasse. Bisogna pagarlo, poi se uno è povero, si darà il pane a chi è povero.

il Parlamento europeo abbia avuto un tempo molto lungo per approvare questa direttiva. Ci sono voluti anni, perché quelli che contrastano sono potentissimi. Badate che la lotta non è affatto finita.

critico verso l'Europa, che pure penso debba essere un grande spazio comune, anzi ci manda una direttiva importante che dobbiamo recepire insieme a tante altre cose di cui non parlerò e di cui parleranno altri colleghi, a proposito della legge europea) ha annullato la multa. Ho letto che la Commissione europea legge europea) ha annullato la multa. Ho letto che la Commissione europea ha fatto ricorso, non voglio accusare di niente nessuno, ma chi deve pagare 14 miliardi di euro il modo per trovare una giustizia compiacente lo quindi far sì che tutto questo progresso che oggi la tecnologia ci offre non ammazzi il resto, non desertifichi l'editoria, la letteratura, la musica, gli autori, la creatività, il pensiero. Quindi è giusto che siano tassati, che paghino il dovuto, che paghino i diritti d'autore

via *web.* È ovvio, è normale. Oggi, attraverso un oggetto come uno *smartphone* guardiamo la televisione o un film, anche se è meglio guardarlo in una sala cinematografica e non su un microschermo, perché anche la fruizione dell'opera nella sua dimensione è consigliabile. Si può fare di tutto, anche leggere un giornale, però è giusto che in qualche modo

di Rete 4 e di quell'altra rete, che sono proprio dei granelli di polvere nel mondo. Oggi ci sono potentati che finiscono per controllare la conoscenza e l'informazione, perché decidono quali film si producono, quali mercati aggredire,

ma proprio della difesa della creatività, per evitare che poi non ci sia nessun fornaio a fare il pane della cultura, del giornalismo, della letteratura, del cinema che poi, ridotto sul lastrico, non può produrre un film perché deve fare un'opera d'arte, perché purtroppo ci vogliono i mezzi. In conclusione,

ci fosse stato Guglielmo Marconi e qualcun altro non ci sarebbe stato nemmeno Internet e tutto il resto), ci sia un po' di equità. La norma in discussione contiene un principio importante, speriamo che venga attuato al più presto in Italia perché serviranno altri provvedimenti

siamo oggi chiamati a esaminare un provvedimento che da sempre è stato colpevolmente sottovalutato, ma che in realtà riveste un ruolo fondamentale per la vita della Nazione: la legge di delegazione europea. La legge di delegazione europea è costituita da una moltitudine di deleghe legislative che il Parlamento cede al Governo al fine di adeguare l'impianto normativo nazionale alle nuove disposizioni comunitarie. Anche quest'anno sono tante le aree in cui si interviene, dalla salute all'ambiente, dalla cybersicurezza alla finanza. Milioni di nostri concittadini dovranno quindi fare i conti con queste nuove norme. Considerando l'importanza di queste leggi, auspico la celere individuazione di modelli che rendano possibile anticipare *ex ante* l'impatto di tale legislazione sul tessuto socio-economico. Spesso infatti subiamo provvedimenti che penalizzano i nostri imprenditori a tutto vantaggio di quelli di Paesi meglio strutturati nella pratica dell'opera di *lobbying* presso le istituzioni europee. Dobbiamo invece imparare a essere molto più preparati su provvedimenti legislativi che sono il *trait d'union* tra Bruxelles e Roma. Provando ad entrare nel dettaglio di questo che, come dicevo poc'anzi, è un provvedimento estremamente complesso ma che interessa diversi ambiti della vita dei nostri cittadini, è necessario prima di ogni cosa fare un passaggio sulle diverse direttive europee che il nostro Paese si accinge a recepire. Su ogni argomento Forza Italia ha provato a dare il suo contributo per un migliore adeguamento delle direttive europee al tessuto legislativo nazionale, tenendo conto delle peculiarità del nostro Paese e per fare in modo che non impattassero in maniera estranea sulla vita quotidiana degli italiani. Devo dire - permettetemi questa piccola digressione - che il dibattito in Commissione è stato sereno, collaborativo e per questo mi sento di ringraziare tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione e il relatore, senatore Pittella, per aver superato gli steccati partitici e aver provato a trovare una giusta sintesi tra le varie posizioni. Probabilmente la complessità dell'atto e la percezione, ovviamente errata, che esso non impatti direttamente sulle politiche nazionali, ha fatto sì che non ci fossero le pressioni esterne che spesso e volentieri hanno incagliato i lavori parlamentari. Detto questo, rientro nel merito del provvedimento citando solo alcuni aspetti su cui abbiamo inciso in maniera significativa. Ad esempio, per ciò che riguarda il settore delle comunicazioni, sia la tutela degli utenti, sia la tutela del diritto d'autore costituiscono un nodo fondamentale per la normativa. Per quanto Forza Italia si sia sempre dimostrata pronta a sostenere il progresso, lo sviluppo e la semplificazione delle nuove tecnologie per la comunicazione, dobbiamo però tutelare con attenzione i diritti dei produttori, ma anche quelli dei consumatori. In questa direzione abbiamo presentato una serie di emendamenti e di ordini del giorno che sono stati accolti, magari riformulati dalla maggioranza - questo sì - affinché nelle deleghe si imponga una maggiore attenzione alla garanzia dei prodotti delle nostre aziende di comunicazione. Manca garantire i singoli artisti, come diceva prima il collega Gasparri, che vedono spesso compromesso il loro diritto di compenso dalle grandi multinazionali extraeuropee dello *streaming* e della diffusione. Altro tema di particolare rilievo su cui abbiamo provato a dare il nostro contributo è quello sullo sviluppo delle energie rinnovabili, un argomento anche questo che sembra forse lontano dai cittadini, ma che in realtà ha un impatto diretto e forte sulle loro vite e sul loro portafogli. Le aziende del settore elettrico rappresentano una leva strategica fondamentale a supporto del rilancio dell'economia del Paese e, secondo il piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il nostro Paese dovrà raggiungere, nel 2030, il 30 per cento di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi. Per il solo settore elettrico, questo *target* si tradurrebbe in un valore pari a oltre il 55 per cento di fonti rinnovabili rispetto ai consumi interni lordi di energia elettrica previsti. Si tratta di una sfida sicuramente ambiziosa per la quale le fonti rinnovabili saranno chiamate a ricoprire un ruolo primario nel mercato elettrico e per conseguire un simile sviluppo dovranno essere previste iniziative che contemplino anche investimenti per rinnovare, e in alcuni casi mantenere in efficienza, gli impianti esistenti. In quest'ottica è imprescindibile superare le barriere, anche normative, che ostacolano il pieno sviluppo delle fonti di energia rinnovabili ed è in questa direzione che dovranno andare le deleghe che il Governo dovrà affrontare il più presto possibile. C'è poi una modifica di cui siamo particolarmente orgogliosi e che è diventata parte integrante del testo che ci apprestiamo a votare: la collega senatrice Rizzotti ha infatti presentato un emendamento per inserire nel novero dei farmaci veterinari prescrivibili in modalità elettronica anche quelli ad azione stupefacente o psicotropa, come già avviene per lo stesso tipo di medicinali in campo umano. Anche questo sembra un intervento lontano dalla vita quotidiana ma l'emergenza Covid ha dimostrato come la dematerializzazione delle ricette mediche sia utile e quanto la tracciabilità e la reperibilità di informazioni relative alla sanità pubblica, e quindi anche a quella animale (perché tutti abbiamo a cuore la salute degli animali), sia fondamentale per una maggiore tutela dei cittadini. Tanti quindi gli ambiti di intervento di questo provvedimento, un provvedimento che dovrebbe dare l'esatta misura di quanto l'Europa e i suoi Stati membri dovrebbero collaborare per un uno sviluppo davvero consolidato e comune. Non posso quindi non fare una breve riflessione sullo stato delle cose rispetto ai rapporti tra il nostro Paese e l'Unione europea ed è impossibile non partire purtroppo dalla tragedia del Covid-19 e dal terribile impatto che questa pandemia ha avuto sulla nostra società e sulla nostra economia. La risposta comunitaria è stata inizialmente balbettante, forse a causa di un'estrema sottovalutazione del problema: l'episodio di egoismo nazionale, con il blocco del materiale alla frontiera, o la lentezza con cui si sono messi in campo gli strumenti necessari ad uscire dall'emergenza hanno fatto - ahimè - vacillare pesantemente in questa prima fase le fondamenta stessa dell'istituto comunitario. Eppure proprio questa legge di delegazione europea, con le sue direttive da recepire e le sue deleghe da assegnare ci dimostra che lo scopo principale dell'Unione è quello di creare percorsi comuni che possano aiutare tutti gli Stati a progredire in maniera sincronica sulla strada dello sviluppo economico, sociale e culturale. Il problema quindi non è l'Europa in sé, ma è l'uso che singoli Stati fanno degli strumenti che l'Europa mette loro a disposizione. Permettetemi quindi in conclusione di fare una sorta di appello al Governo, a cui oggi consegniamo una serie di deleghe che gli consentiranno di legiferare sugli argomenti più disparati, ma al contempo, sempre in tema europeo, ha la grande responsabilità di stilare progetti attrattivi e funzionali per usufruire dei fondi del *recovery fund*. Con il programma Next generation EU l'Europa ha l'ambizione di trasformare le macerie lasciate dal Covid-19 in un'opportunità per ricostruire un Continente più efficiente, più moderno e più *green*, un'Europa dei diritti e delle opportunità; un'area in cui la libertà economica e sociale permetta a tutti di costruirsi un futuro di speranza e di successo. Ma l'Europa, tanto quando sbaglia, tanto quando fa la cosa giusta, non è sola; è una comunità. Il mio appello al Governo va proprio in questo senso. Non fate tutto da soli per favore, non gestite questi fondi da soli. Si crei un percorso di collaborazione, perché non è accettabile che il *recovery plan* italiano sia rappresentato da poche pagine scritte fra di voi e senza coinvolgimento alcuno del Parlamento e della società civile. Non è così che sfrutteremo la straordinaria opportunità che l'Europa ci offre e non è così che cambieremo il volto dell'Italia. Forza Italia ha da subito manifestato la propria assoluta e sincera disponibilità a dare una mano. C'è bisogno di unità di intenti e di superare gli steccati ideologici per riuscire a portare l'Italia fuori dalla situazione in cui ci troviamo. Con questo provvedimento in Commissione abbiamo dimostrato che è possibile farlo. Ora sta al Governo accettare la sfida e lasciare da parte le divergenze spicciole per perseguire obiettivi comuni. Non lo chiedo io, lo chiede a gran forza il Paese. Signor Presidente, potremmo argomentare in diverse maniere, andando a vedere - come ha detto prima anche il relatore - gli emendamenti o i singoli articoli di questo dispositivo di legge o la stessa relazione di partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Ma mi limiterò ad alcuni elementi, tre in particolare, che credo siano stati abbastanza emblematici di come purtroppo la maggioranza di Governo, per l'ennesima volta, ha utilizzato male uno strumento così importante come la legge di delegazione europea, banalizzando alcune situazioni che invece necessitano di grande considerazione, a nostro avviso, oppure semplicemente per partito preso, dicendo di no, perché a proporre queste cose era l'opposizione. Quella stessa opposizione che prepara emendamenti e li propone e non mi si venga a dire che poi si deve anche votare a favore, perché qualche emendamento viene accolto. Questo è un provvedimento estremamente ampio. Quello che abbiamo chiesto innanzitutto alla Commissione, ovvero alla maggioranza, è che ci fosse consapevolezza di che cosa vuol dire acquisire, a normativa italiana, disposizioni europee che portano poi costi sulle nostre imprese e costi sulle nostre attività produttive, tanto più in un momento grave come quello che stiamo vivendo di crisi economica. Tutto questo, Presidente, è stato

«Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo assicura che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle amministrazioni centrali, sulle autorità amministrative indipendenti, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano: il meno gravosi possibile; b) commisurati all'obiettivo da conseguire; c) adeguatamente attenuati attraverso la concessione di contributi o detrazioni». Un concetto molto semplice. C'è una normativa europea, questa viene recepita. Bisogna considerare che questa per essere recepita comporta dei costi, che spesso e volentieri mandano le nostre imprese fuori mercato. Allora noi abbiamo fatto una considerazione: si mettano a disposizione, come dicevo, detrazioni e anche contributi diretti, in modo tale che la normativa possa essere recepita velocemente e agevolmente, ma nello stesso tempo si eviti di gravare in maniera determinante, tanto più in una circostanza nella quale la nostra economia è tanto messa a dura prova con questa crisi economica. L'emendamento non è stato recepito da parte della maggioranza. Al limite in questi casi ci si limita all'ordine del giorno o alla raccomandazione che purtroppo - lo dico ancora una volta - troppo inflazionati, hanno perso di qualsiasi significato. Anzi, se c'è una modifica da fare al nostro Regolamento e anche nel rapporto tra Governo e Parlamento, Presidente, sarebbe proprio quella di stabilire che se si prende un impegno, che sia una mozione, un ordine del giorno o una raccomandazione, quando la si prende, lo si fa seriamente e poi se ne deve dare conto.

naso. Questa è la prima questione: è stato sottovalutato completamente l'impatto economico di questa normativa tanto più in una situazione di grave crisi economica. Badate bene; non sto dicendo né bene, né male, sul fatto di recepire la normativa. Dico solo che recepirla senza considerare il costo che essa produce, tanto più in una circostanza come questa, può produrre due effetti, caro relatore: mettiamo i nostri cittadini e le nostre imprese in obbligo di seguire norme che trasgrediranno, perché rispettarle può voler dire andare fuori mercato, oppure che noi stessi alleggeriremo ovviamente la maglia dei controlli, perché altrimenti chiudiamo le nostre imprese, ci troveremo in infrazione e creeremo una condizione paradossale. Abbiamo recepito la norma, ci siamo messi a posto con la forma, ma nella sostanza tutto questo crea un ulteriore problema. Mi soffermo poi su un'altra questione che non è da meno.

non la leggerò tutta, ma per ovvia brevità, vado direttamente in fondo: alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i tempi di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7 la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forze di tali disposizioni. Per questi motivi la Corte, in grande sezione, dichiara e statuisce non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni. In secondo luogo stabilisce che la Repubblica Italiana è condannata alle spese. Presidente, c'è una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 gennaio, che mette nero su bianco che l'Italia sta trasgredendo gli obblighi che ha nel pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e nei tempi stabiliti dalle stesse direttive europee. Lo sapevamo già, ce lo dicono oggi con sentenza. A fronte di questo, essendo il provvedimento in transito in Senato, presentiamo un emendamento estremamente semplice

«Al fine di giungere al recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di giustizia dell'Unione europea - Grande Sezione, nella causa per "Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni

adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione; *c)* determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora

presenza del sottosegretario Castoldi, in Commissione, la mia domanda è stata: «Perché il Governo esprime parere contrario?». Non c'è stata alcuna risposta. Aveva davanti uno *speech* su cui era scritto parere contrario: o non sapeva cosa c'era scritto

Questa è la considerazione che oggi il Governo sta dando ai debiti della pubblica amministrazione. Ritengo che tutto ciò sia quanto meno inaccettabile. *(Applausi)*. A fronte di questo dico solo che stiamo facendo e state facendo un disastro: se in questo momento si danno soldi alle imprese e si lasciano i soldi nelle casse della pubblica amministrazione, non pagando,

fatto di natura emotiva, prima di entrare nel discorso tecnico e di merito. Il fatto è questo. Per una coincidenza questo fine settimana sarò a Ventotene con un gruppo di ragazzi e di ragazze del mio territorio ad approfondire i temi dell'Europa e a ragionare su quelle origini. Proviamo per un secondo a pensare, noi che siamo in Aula, se Altiero Spinelli oggi entrasse da quella porta e sapesse che il Parlamento italiano, il Senato della Repubblica in particolare, sta discutendo nel merito di alcuni provvedimenti che devono essere recepiti da tutti i Parlamenti nazionali e da tutti i Governi nazionali e che provano a diventare una legislazione positiva per far compiere dei passi avanti ai cittadini europei rispetto al futuro della loro vita. Vedete, quando noi parliamo di sogno europeo e quando usiamo parola - sogno - qualche volta può sembrare qualcosa di molto lontano e di molto astratto. Invece il sogno è questo: è quella capacità che hanno gli uomini di immaginare un futuro che non c'è in quel momento e quella tenacia, quell'ostinazione, quella forza e quella capacità creativa di realizzarlo. Da un gruppo di persone esiliate per un confino politico su una piccola isola del Mediterraneo nacque un sogno che oggi non è neanche lontanamente realizzato, ma in cui alcune delle conseguenze si misurano nei fatti concreti, nella vita quotidiana di tutte le persone, ogni giorno che passa. Ho usato una parola, creatività: questa è una delle conseguenze più importanti di questa direttiva. direttiva. Ciò di cui hanno parlato molto bene la collega Fedeli e altri colleghi che sono intervenuti in Assemblea e su cui si è concentrato molto il lavoro della Commissione, ossia il recepimento di quella parte cosiddetta sul *copyright*, io la definirei come la tutela del lavoro creativo, la tutela dei diritti dei lavoratori della creatività. Noi non abbiamo niente di antimoderno, siamo assolutamente convinti che le tecnologie siano una grande occasione per il progresso personale. Tuttavia non possiamo pensare che qualcuno

svolto; questo è tutt'altro che moderno, ma è qualcosa di straordinariamente antico, che conosciamo, vecchio come l'uomo, ed è uno dei motivi per cui nasce la politica. La politica nasce esattamente per costruire delle norme efficaci e positive che redistribuiscano i redditi e soprattutto diano a chi crea, a chi lavora, a chi produce col proprio tempo, con la propria fatica, con la propria energia quanto gli spetta, soprattutto a chi è più debole. È quindi oggi evidente che, di fronte a qualcuno che è molto forte e che in realtà costruisce e realizza molto poco e però guadagna molto sul lavoro e sulla fatica di chi è spesso molto debole, serve un organismo sufficientemente forte, sufficientemente capace e necessariamente politico, che restituisca quel valore a chi lo ha realizzato. Questo è il senso dell'importantissimo punto di equilibrio trovato al Parlamento europeo. sottolineo queste parole, perché il nodo è proprio quello: la politica è questo, è costruire un punto di equilibrio tra culture diverse, tra Paesi diversi, tra Stati che hanno al loro interno culture diverse anche su questi temi, e trovare il modo per renderlo efficace.

figli una cultura europea - tuteliamo molto meglio il diritto d'autore e lo restituiamo giustamente agli autori americani, ma dall'altra parte dell'oceano non ci torna neanche lontanamente la stessa cifra, perché, in una logica un po' diversa, in cui governa molto il più forte (perché c'è un'idea malintesa, a mio parere, di libertà della contrattazione e dei diritti), solo i grandi autori riescono a tutelare la loro creatività e tutti i piccoli autori non vengono tutelati; e tanti di questi sono anche i nostri autori. L'altro tema che voglio solo sfiorare e che è stato in parte citato è quello delle energie rinnovabili.

creatività sia all'origine di questa capacità innovativa; e poi perché, ancora una volta, viene dall'Europa una spinta, che viene rafforzata proprio in queste ore, con il voto che il Parlamento europeo sta realizzando sulla legge sul clima, per cui noi siamo al recepimento di alcune norme costruite nel passato e nel frattempo quel luogo di elaborazione prosegue

vengono stimolate dalle norme che spingono a fare meglio, perché la capacità imprenditoriale è proprio questo: non ha mai niente a che vedere con la conservazione dello *status quo*, ma è la capacità di immaginare un'idea

competere - anche se è una parola che non amo molto - nel mercato globale, invece di difendere le proprie posizioni del passato. Sono convinto che le imprese italiane abbiano solo da guadagnare da una normativa comunitaria

dare spazio a nuovi lavori e a nuove capacità di impresa che pensino a un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze di futuro che la situazione del nostro pianeta ci impone.

facendo tesoro di ciò che grandi italiani come Altiero Spinelli hanno saputo realizzare.

si dichiari immediatamente, come abbiamo già chiesto nella giornata di lunedì, lo stato di emergenza per la terribile calamità alluvionale che ha colpito il Piemonte. Ieri il governatore Cirio è stato dal ministro dell'interno Lamorgese per comunicare una prima stima

secondo appello che faccio subito oggi è per quei 18 pescatori italiani che sono ancora prigionieri in Libia senza un'accusa precisa. Oggi i familiari hanno protestato davanti a Montecitorio. Il Governo, che così tanto si è dato da fare in questi giorni per i migranti, dimostri almeno un po' di dignità per i cittadini italiani e riporti a casa i nostri ragazzi! È il momento della responsabilità: lo dimostrino il Presidente del Consiglio, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno.

Certamente parliamo dell'importante tematica delle pratiche commerciali sleali, che riguardano soprattutto il mondo agroalimentare, ma non solo. L'Italia ha già provveduto a disciplinarle con l'articolo 62, con l'articolo 62, che prevede una regolamentazione molto avanzata dei rapporti commerciali, relativa alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari, con punti di forza ulteriori rispetto alla stessa direttiva europea. Rimangono, però, alcuni

le pratiche europee sono difficili da inquadrare a livello di violazione dell'attuale legislazione in materia di concorrenza. Dato che gli strumenti messi a disposizione dalla normativa nazionale ed europea sono efficaci soltanto a contrastare alcune forme di comportamenti concorrenziali, con il recepimento della direttiva 2019/633 si sarebbe potuto intervenire proprio su questo aspetto. In realtà, il testo, così come modificato in Commissione, rischia invece di inficiare quanto di positivo è stato fino ad oggi compiuto dal nostro Paese per riuscire a individuare la presenza, all'interno di una filiera economica, di un'eventuale pratica sleale. Affidare a due organi diversi come l'Icqrf e l'AGCM significa rendere inefficace un intervento sanzionatorio nei confronti di eventuali trasgressori. Potrebbero infatti nascere una serie di contenziosi e ricorsi per mancanza di competenza dell'autorità coinvolta, che avrebbero l'effetto di ingessare l'attuale assetto normativo e di lasciar continuare la pratica sleale senza alcun tipo di provvedimento. Un aspetto che necessariamente dev'essere migliorato è quello dell'efficienza della filiera agroalimentare; bisogna rivedere alcune dinamiche. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva aperto, in virtù delle competenze attribuitele, due indagini sul settore lattiero-caseario riguardanti la dinamica della formazione dei prezzi della filiera. La necessità dell'indagine risiedeva nel fatto che, oggi più che mai, le dinamiche che regolano la formazione dei prezzi sono poco trasparenti e le informazioni sono molto frammentate; il latte ne è un esempio, come la zootecnia. Di qui ricade poi che, nella suddivisione corretta dei margini e dei ricavi all'interno della filiera, i più penalizzati sono i produttori primari, gli agricoltori e le nostre stalle: il prezzo del latte oggi è di 35 centesimi, a fronte di un costo, per chi lavora, si alza al mattino alle 4 e fino alla sera è preoccupato e lavora in stalla, di 0,40 centesimi; c'è una perdita secca su questi prodotti, ma non solo. C'è anche sulla zootecnia, che sulla parte carne, ha problematiche enormi e costi di produzione elevati, a fronte di una filiera che poi non riporta indietro le necessarie e dovute spettanze a livello di redditività. Abbiamo davanti a noi una grande opportunità, che ci viene data dalle risorse del *recovery fund*, per dare competitività alla filiera agroalimentare italiana. Il Ministro, nel corso dell'audizione che abbiamo svolto presso la nostra Commissione sulle politiche agroalimentari, ci ha parlato di un parco progetti pari a 17 miliardi di risorse economiche. Sappiamo che la filiera agroalimentare nel periodo dell'emergenza è stata straordinariamente importante ed è riuscita a superare anche il *lockdown* delle altre imprese, attività e filiere ad essa collegate; parliamo della parte automazione, delle macchine e delle attrezzature necessarie. Ma questo ruolo strategico non si rivela poi nei fatti, perché oggi si parla di poche risorse, circa un miliardo di euro al settore agroalimentare, rispetto ai 17 necessari. Abbiamo bisogno di sapere quali sono le risorse certe, i tempi di applicazione e soprattutto chi dovrà determinarne l'erogazione. Non può farlo il Governo da solo, ma deve coinvolgere necessariamente le Regioni, perché si tratta di un progetto importante di rilancio di un settore straordinario del nostro Paese. Vi ricordo che la Politica agricola comunitaria (PAC) ha subito un taglio di circa 34 miliardi di euro. Le ripercussioni sono da subito evidenti a livello nazionale: è previsto un taglio di 370 milioni già nel 2021, il 4 per cento in meno sui piani di sviluppo rurale e 15 per cento in meno sui pagamenti diretti agli agricoltori. Parliamo di un settore, l'agroalimentare, che vale 540 miliardi, con 119 miliardi di valore aggiunto, 3,6 milioni di occupati, 2,1 milioni imprese e quasi 50 miliardi di euro di *export*. Perciò chiediamo

Signor Presidente, consenta anche a me di ringraziare i relatori, e in particolare il senatore Pittella, per il lavoro svolto durante l'esame del disegno di legge di delegazione europea, ma anche il sottosegretario Agea, che è stata con noi

alle tante audizioni che abbiamo svolto con i rappresentanti e i diversi portatori di interessi diffusi, oltre che al dibattito che si è svolto nella Commissione Il disegno di legge in esame è un provvedimento importante, com'è stato già ricordato, perché contribuisce in maniera significativa al processo di avvicinamento delle normative

rimane fattibile, di un'Europa unita anche politicamente, oltre che dal punto di vista dell'avvicinamento dei sistemi economici e, in futuro, speriamo anche di quelli sociali. è un disegno di legge su cui l'Italia si gioca un pezzo della propria credibilità, grazie al contributo offerto alla riduzione del numero delle procedure di infrazione e per evitare l'apertura di nuovo contezioso, anche se, in questo momento, la nostra la nostra credibilità si giocherà soprattutto sulla capacità che sapremo mettere in campo nella predisposizione del Piano nazionale di rilancio e resilienza, per l'impiego delle importanti risorse di Next generation EU, un lavoro parallelo all'esame della legge di delegazione europea, che a volte ha fatto anche sembrare superato l'esame dei provvedimenti contenuti nel disegno di legge in oggetto, ma che invece dobbiamo ritenere complementare serie di articoli molto importanti, con i quali si dà attuazione a ben 33 direttive e 14 regolamenti europei. Di particolare interesse per il mio Gruppo l'articolo 3, recante delega per l'attuazione della direttiva del 2018 sui servizi *media* e audiovisivi, mediante modifiche al testo unico in vigore, che è del 2005, per aprire la strada a un contesto normativo più equo per il settore audiovisivo, stato detto, compresi i servizi *on demand* e la piattaforma di condivisione video, per una maggior tutela dei minori, nello specifico, per la lotta contro l'incitamento all'odio, per la promozione delle produzioni europee e a garanzia dell'indipendenza dell'Autorità di regolamentazione del settore. Il nostro impegno, in particolare, si è concentrato nel chiedere che i fornitori dei servizi *media*, comprese le piattaforme *social*, forniscano informazioni in merito a ogni contenuto che possa nuocere allo sviluppo psicofisico dei minori, compreso il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, nonché misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi, al fine di alterare lo scambio di opinioni, generare allarmi e trarre vantaggio dalla divulgazione di false notizie.

così come l'articolo 4, che contiene un quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi, nonché i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G ad altissima velocità, che è necessario mettere in relazione alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico. Il successivo articolo 5 interviene, inoltre, per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e sulle indicazioni, da parte dei singoli Stati membri, degli obiettivi da raggiungere per il 2030. L'attuazione della direttiva è strettamente connessa con gli articoli 12 e 19, concernenti entrambi il mercato interno dell'energia. Vi è particolare attenzione alla produzione di energia da fonti rinnovabili secondo il criterio della neutralità tecnologica, nonché il principio di riuso e riciclo legati al processo produttivo di un'economia compiutamente circolare, con la promozione di fonti rinnovabili e non inquinanti sia per l'autoconsumo, sia di comunità, con particolare attenzione al trasporto pubblico e, in prospettiva, anche a quello aereo (il riferimento è ai biocarburanti). L'auspicio è che proprio gli enti più prossimi al territorio (quindi i Comuni) possano pianificare un minor consumo di aree e la riconversione di quelle non utilizzate, collegandole all'installazione di nuovi impianti verso uno sviluppo sostenibile, *smart* e intelligente, in linea con il settimo Programma d'azione per l'ambiente, nella consapevolezza che proprio la tutela della salute umana deve fare i conti con la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto al cambiamento climatico, come abbiamo ben appreso anche a causa delle devastazioni di questi ultimi giorni. L'articolo 6 interviene in materia di mercato interno per conferire alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci. L'articolo 7 detta principi in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare e introduce quindi elementi di maggior trasparenza, a beneficio della stessa filiera e dei consumatori finali. Particolarmente importanti sono le norme successive sull'esercizio del diritto d'autore, già richiamato da quest'Assemblea, e i diritti connessi, volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di trasmissioni *online* e la tutela del diritto d'autore nel mercato unico digitale. I successivi articoli intervengono in materia di enti finanziari e creditizi, di imprese di investimento e di accesso al credito delle piccole e medie imprese, ma anche di cybersicurezza e sicurezza informatica.

per la valutazione preventiva delle proposte di legge della Commissione europea, nell'ambito di quel dialogo politico che veda maggiormente protagonista il nostro Paese nella costruzione dell'ordinamento giuridico europeo e, quindi, nel processo di avvicinamento dei Paesi membri, ripensando anche a una più stretta collaborazione con le Regioni, anch'esse loro chiamate a dare attuazione agli atti normativi europei nelle materie di loro competenza. È un lavoro importante, quello della partecipazione del nostro Paese alla costruzione europea, che può vederci quindi protagonisti, nell'interesse degli italiani e di un'Europa che venga percepita sempre più utile e vicina ai bisogni sia dei cittadini, sia delle imprese. I temi trattati nel disegno di legge di delegazione europea sono complementari e in stretta relazione con l'obiettivo della transizione verso un'economia verde e neutrale dal punto di vista dell'impatto ambientale al 2050 verso un'economia digitale, coerente quindi con l'importante lavoro di costruzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sta impegnando Governo e Parlamento in questi giorni, in attesa del Regolamento della Commissione, in vista anche del termine dell'aprile 2021,

i risultati raggiunti nel Consiglio europeo del luglio scorso, per approntare strumenti utili a superare finalmente la grave crisi generata dalla pandemia Covid e le gravi conseguenze economiche e sociali prodotte.

il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato questa norma, credo che tutti coloro che seguono il mondo agricolo e hanno a cuore i temi della qualità, della sicurezza, della sostenibilità sociale, Grazie Il percorso che ci viene adesso affidato, dopo l'approvazione, è quello di mettere il Governo nelle condizioni di emanare i decreti legislativi attuativi per dare vita nel concreto a ciò che contiene l'importante direttiva n. 633 del 2019. È importante perché si mette un punto fermo e si attivano riferimenti normativi e strumenti per incidere sul funzionamento di un sistema di relazioni commerciali in agricoltura che ormai in moltissimi casi è di fatto patogenico, sbagliato e da ripensare. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di pratiche sleali, che posso riassumere con alcuni esempi: ritardi nei pagamenti ben oltre quanto previsto dagli accordi commerciali; modifiche unilaterali retroattive dei contratti; cancellazione di ordine senza preventivo; pagamenti tagliando, a detta dell'acquirente, i prodotti deteriorati senza possibilità di contraddittorio; imposizione di pagamenti di servizi e iniziative non correlati alla vendita del prodotto agricolo da parte di soggetti più forti sul piano commerciale; rifiuto di sottoscrivere contratti scritti; abuso di informazioni confidenziali;

da un dato che può sembrare banale, ma in quelle settimane c'è stata una maxi fusione di centrali di acquisto da parte della centrale Carrefour e della centrale Tesco, che hanno creato un raggruppamento d'acquisto a livello europeo che supera i 150 miliardi di euro di fatturato. Capite che per il mondo agricolo e per quello della trasformazione di prodotti agricoli rapportarsi con un colosso d'acquisto che ha un valore

decine di fornitori di presentare offerte di prodotti con capitolato *a latere*; poi, prendere il prodotto con il prezzo più basso e il capitolato più vantaggioso e su questo chiedere a tutti

che ci sia la necessità di una grande attenzione alle dinamiche di mercato, ma questo deve avvenire in un quadro di regole certe e ferme, che siano forti, perché la libertà di mercato senza regole o con regole deboli o inapplicabili è di fatto una sorta di *far west*, e in queste situazioni il più debole paga il conto di tutti.

e in questa delega che diamo al Governo includiamo quella a ricoordinare tutto il quadro normativo con l'articolo 62. Credo che questa sia una cosa assolutamente ben fatta. Dobbiamo essere riconoscenti

un'azione che può essere veramente utile a tutto il Paese e non soltanto all'agricoltura. Penso che tutti vogliamo un'agricoltura che non sia piegata e sfruttata e che non abbia sacche che, con un'idea impropria di recupero di competitività, sfruttino i lavoratori, violentino l'ambiente o ignorino le norme elementari di sicurezza. Non vogliamo che imprese più grandi o grandi gruppi della grande distribuzione possano fare utili ai danni di imprese più piccole o meno capaci di condurre; quantomeno, vogliamo intervenire per ridurre tutto questo. Non siamo sognatori, ma abbiamo la convinzione che il mercato debba essere regolato, per permettere a tutti gli attori che operano correttamente,

a prevaricazione o abusi di potere. Questa norma ci mette in mano gli strumenti per andare con forza in tale direzione.

nel merito e nel metodo. Nel merito, ovviamente, per l'importanza della legge di delegazione e per il quadro in cui viene approvata, ma anche nel metodo, perché finalmente quest'Assemblea tornerà a votare gli emendamenti, e quindi un provvedimento senza la fiducia (il che dovrebbe essere la norma, ma è diventata l'eccezione). A maggior ragione, quindi, è importante - e ringrazio i relatori per l'attenzione - che ci sia una discussione generale in cui si possa illustrare l'argomento e anche gli emendamenti che responsabilmente, come abbiamo presentato. Quello che chiedevamo e che purtroppo non c'è stato - lo ricordava il senatore Candiani - era una visione complessiva, d'insieme. Tuttavia, abbiamo cercato comunque di migliorare il testo e su questo abbiamo preso atto della disponibilità dei relatori. Come abbiamo detto più volte (valeva per il decreto semplificazioni, è valso ieri nella discussione sulle linee guida sul piano di rilancio e resilienza), c'è sempre qualcosa da aggiungere: lì siamo al limite, perché, su 38 pagine, una è sull'ambiente, mentre il parere della Commissione ambiente sarà di 30 pagine, quasi quanto l'atto principale. Questo per dire che si può sempre migliorare e aggiungere qualcosa e farò tre esempi per quanto riguarda il provvedimento che ci accingiamo a votare: uno riguardo all'articolo 5; uno riguardo all'articolo 6 e uno riguardo a sarà l'articolo 22, visto il nuovo ordine nel testo che arriva in Aula. L'articolo 5, sulle energie da fonte rinnovabile, va benissimo, è ottimo; anzi, dalla Commissione è uscito particolarmente modificato il testo base, con molte aggiunte. Si è pensato a tutto: a dove collocare i pannelli fotovoltaici e alla questione delle ex discariche (ne abbiamo parlato e, anche come Gruppo Lega, abbiamo presentato emendamenti su questo). Manca l'ultimo metro:

ma se ciò comunque produce rifiuti, non pensare anche a questo aspetto e non chiedere al Governo di recepire la direttiva europea in tale direzione (ce n'è una) è sicuramente una mancanza che c'è modo di colmare, per avere anche l'ultimo metro e chiudere

sta salvando dai contagi *(Applausi)*. Pertanto, un attacco ideologico alla plastica come materiale è dannoso, oltre che assolutamente ingiustificato.

che siano assicurate definizioni chiare al fine di delimitare correttamente il perimetro d'applicazione delle misure, soprattutto per i contenitori per alimenti. Dire che si debbano individuare i meccanismi volti ad assicurare un passaggio graduale, che consenta la riconversione, è fondamentale: in parte, come Lega lo abbiamo fatto nella manovra finanziaria approvata nel dicembre 2018 (mi sembra fosse il comma 652 che proponemmo allora). Perché dobbiamo essere sempre i primi della classe? Se l'Europa ci dà dei tempi, perché non dobbiamo utilizzarli tutti? È

avevamo chiesto, come il collega Candiani ha ribadito più volte, l'impegno affinché l'adeguamento della normativa vigente sia fatto evitando aggravi procedurali ed economici eccessivi per le aziende.

è una facoltà per gli Stati: la Germania l'ha colta al volo, noi aspettiamo da un anno e mezzo. L'impegno è rivolto al Governo e c'è una volontà unanime, credo sia politica sia del tessuto economico, di recepire

il 14 agosto del 2018, come tutti sapete, è crollato il ponte Morandi a Genova. Nell'immediatezza dell'evento, due giorni dopo, per l'esattezza, il Ministero inviò una lettera di contestazione di addebito all'Aspi, la società che gestiva la concessione. Da allora sono passati più di due anni e il procedimento amministrativo non si è ancora concluso. Il 15 luglio 2020, però, il Consiglio dei ministri ha emanato un comunicato in cui ha affermato il raggiungimento di un'intesa transattiva. In particolare, la questione centrale di quest'intesa sarebbe stata l'immediata fuoriuscita da Aspi di Atlantia e dei Benetton, con passaggio del controllo a un soggetto a partecipazione statale.

perché qualcosa, dopo due anni, si deve pur fare. Lo si deve ai parenti delle 43 vittime del disastro, ad una città e ad un Paese che sono rimasti attoniti,

Signor Presidente, oggi in quest'Aula vorrei ricordare e commemorare il sacrificio del sottufficiale

Lo vogliamo onorare in quest'Aula perché, oltre ad aver compiuto il suo dovere, era un uomo, un ragazzo, che effettivamente era testimonianza di gentilezza e di generosità nella sua vita. Spero che venga fatta chiarezza sulle dinamiche della sua morte, in modo che la famiglia possa trovare totale conforto e spiegazione. Ad ogni modo, mi piace ricordarlo come fa la famiglia: eroe da vivo, perché effettivamente eroi si può essere una volta soltanto; uomini, però, bisogna esserlo ogni giorno e lui lo era, con grandezza.

tutti coloro che si sacrificano nell'esercizio del loro dovere. Grazie veramente di cuore.

ai manifesti di minaccia contro il questore De Matteis, il prefetto Palomba, il dirigente della Digos Ambra e alcuni magistrati, tra cui il procuratore generale Saluzzo; alla busta contenente due proiettili 9x21, giudice Bonu rea solo di aver negato misure alternative alla detenzione per la portavoce del Movimento No TAV Dana Lauriola: i volantini parlano di «mafia del TAV in questura, prefettura e tribunale». Sono state fermate due persone di

Il fatto che per gli inquirenti i manifesti raffiguranti il presidente Cirio e quelli sui magistrati non siano collegabili è dal mio punto di vista oltremodo preoccupante. Il tutto non deve essere preso come uno scherzo goliardico e non deve essere sottovalutato, vista anche la non tenera età dei due arrestati. Questa è l'ennesima conferma che la TAV è solo una scusa. Questi signori vogliono sfidare le istituzioni e con esse lo Stato. Come personalmente già denunciato in più occasioni in quest'Aula, è ora che le istituzioni ne prendano atto e diano dimostrazione di contrasto fermo a questo tipo di atteggiamento. È ora che le forze politiche che compongono il Governo, specialmente una, prendano le distanze e condannino fermamente e ufficialmente i contestatori no TAV che, come dimostrato dai fatti, non c'entrano nulla con i valligiani, ma molto c'entrano con gli anarco-insurrezionalisti. È ora che il ministro De Micheli dia il via alla partenza dei lavori delle nicchie sul versante italiano, dal momento che in Francia i lavori per l'Alta velocità non si sono mai fermati. Torino e l'Italia hanno già vissuto un periodo di terrore negli anni Settanta e i torinesi sinceramente non meritano di ripiombare in questo incubo.

Signor Presidente, utilizzo questi tre minuti perché, anche se abbiamo terminato la discussione sul decreto agosto, ci sono impegni che è opportuno ricordare in quest'Aula,

di bilancio che le Camere affronteranno a breve. Le questioni sono tre. La prima riguarda la partita - chiamiamola così - del turismo,

C'era la possibilità di individuare un percorso per le Regioni del Centro Italia, in modo particolare quelle colpite dal sisma, e si poteva magari fare un'operazione come

pur essendo tutta l'Umbria una città d'arte, dove ci siamo anche visti con la senatrice Pavanelli), proprio perché sono aree particolarmente colpite e provate. Stesso ragionamento per la decontribuzione la decontribuzione dagli oneri sul lavoro dipendente: anche in questo caso si potevano individuare delle aree, sempre comprese nelle quattro Regioni colpite dal sisma dell'agosto del 2016,

come raccomandazione. Voglio quindi ora ricordare in quest'Aula, alla presenza anche di chi aveva seguito queste vicende, che c'è la volontà di tutte le forze politiche

gli emendamenti e gli impegni che si erano assunti, la problematica relativa all'estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza

ogni momento del dibattito parlamentare debba essere utilizzato per ricordare questi impegni che si trascinano di decreto in decreto e che il Governo deve assumere. **Atti e documenti,